Comunico che in data 2 luglio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare:* «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»

hanno evidenza. Già nell'articolo 1 c'è una prima grande risposta al mondo dell'agricoltura rispetto alla moratoria sui mutui, tanto richiesta dalle aziende che avevano subito un 20 per cento di calo di fatturato o del 30 per cento della produzione, aggiunto poi in Commissione, che consente loro di avere una boccata di ossigeno in un momento difficile. Non ci si è limitati però solamente a questo. Ci sono oltre 21 milioni a copertura dei costi per interessi di finanziamenti bancari per le aziende agricole e della pesca;

particolarmente colpite (settore oleario, agrumicolo, lattiero, caseario e ovicaprino) a copertura dei costi di interessi dovuti nel 2023 sui finanziamenti bancari relativi alle OP. un rifinanziamento del fondo delle filiere di 32 milioni; 12 milioni per sostenere la filiera del grano e 20 per affrontare il dramma del granchio blu. E ancora nel 2024 per la ZES unica del Sud; 4 milioni con la nuova istituzione, per volontà e merito del corelatore Bergesio, per sostenere le razze autoctone in via di estinzione o comunque problematiche per allineare l'Italia a ciò che fa già il resto d'Europa, tutelando le proprie produzioni a scapito invece di quelle magari acquisite in altre aree.

Non è un caso il limite al 2025 perché noi auspichiamo che la prossima Commissione europea riesca a legiferare finalmente in maniera moderna su un tema come quello delle TEA, che ha avuto occorre ricordare - anche episodi spiacevoli e sgradevoli, come l'attacco al campo della provincia di Pavia, dove c'è stata la prima sperimentazione a terra,

contro un volere democratico di questo Senato che quasi alla totale unanimità aveva votato per la sperimentazione a terra, ma anche vanificando tanto lavoro dei nostri ricercatori che da anni ci chiedono, insieme alle associazioni agricole, di intervenire sul tema. tema. È stato approvato poi un "emendamento frane" dell'opposizione, presentato nello specifico dalla collega Aurora Floridia, con il quale sono stati inclusi tra gli interventi indennizzabili anche quelli causati alle produzioni agricole ed alle aziende ubicate nei territori alluvionati di Emilia-Romagna, Toscana e Marche dalle frane e da altri eventi alluvionali. A questi interventi abbiamo riservato fino ad 8 milioni. Siamo intervenuti anche sulle spese che i Comuni affrontano per la gestione della Carta dedicata a te,

con l'omicidio del povero bracciante abbandonato sostanzialmente privo di un braccio, che rappresenta una pagina buia non dell'agricoltura, ma di un contesto sociale difficile, che soprattutto

quattro emendamenti dei relatori; uno sugli ammortizzatori sociali, l'altro sul rafforzamento dei controlli per il contrasto all'illegalità e al caporalato; si concede sostanzialmente l'accesso ai dati dell'INPS e alle altre banche dati del personale dell'INAIL, al Comando dei carabinieri a tutela del lavoro e alla Guardia di finanza, con l'assunzione di 403 unità di personale ispettivo INPS e di 111 unità dell'INAIL.

e sul numero susseguente dei loro occupati. C'è poi la banca appalti, alla quale si devono iscrivere tutte le imprese che partecipano a gare dove il committente è impresa agricola. Questo è fondamentale per contrastare il fenomeno delle imprese "senza terra", di quelle imprese che operano in modo irregolare. Qui si stabiliscono anche le regole per la stipula. Ci sono poi tanti altri interventi, come quelli sul kiwi e sulla peronospora, dove gli emendamenti relatori hanno superato di parecchio gli emendamenti dell'opposizione, a dimostrazione che è vero che si può fare sempre di più, ma certe volte si fa molto nei decreti e si può lavorare molto anche in Commissione. Lo dico sulla peronospora, sulla flavescenza dorata, sul bostrico, con 9 milioni dedicati in tre anni al contrasto di queste nuove malattie e di questi nuovi batteri, che insieme alla Xylella flagellano le nostre colture e che sono frutto anche del cambiamento climatico, per il quale probabilmente negli anni precedenti non avevamo un monitoraggio tale da consentire di capire prima ciò che accadeva. C'è l'articolo 4, che disciplina le norme sulle pratiche sleali. C'è l'introduzione del Granaio Italia. C'è la grande partita del divieto del fotovoltaico a terra: basta consumo di suolo agricolo. Abbiamo investito molto sull'agrifotovoltaico, dove l'Europa ci ha concesso ulteriori 800 milioni, oltre al miliardo e 500 milioni già stanziati, ma non ha senso, in un mondo che dovrà produrre di più è meglio, consumare il suolo agricolo. consta di circa 350 milioni di euro, esclusa la parte Ilva, dove c'è naturalmente il prestito di 150 milioni per mettere una pezza all'ennesima situazione di difficoltà. Ciò che attiene all'agricoltura oggi raggiunge e supera i 350 milioni di euro, a dimostrazione di un impegno concreto e serio, che ha avuto non solo nei numeri, ma anche nelle anche nelle manifestazioni di supporto delle aziende agricole, un'ottima evidenza.

l'utilizzo consapevole del suolo agricolo, le pratiche commerciali sleali, la trasparenza dei mercati. Avevamo una situazione drammatica, dove i nostri agricoltori e produttori vanno al mercato senza avere la possibilità di capire quale sarà il prezzo della merce che avranno la possibilità di ottenere a fine mercato. Un po' di chiarezza e di regolarità, soprattutto nell'approccio verso il mercato, ci voleva, responsabilizzando anche qui la struttura mercatale italiana, che è molto forte e si è resa disponibile. Oltre a questo, viene viene istituito un conteggio reale della valorizzazione dei prodotti agricoli, attraverso il percorso dell'individuazione del costo di produzione, sia di quello puntuale che di quello medio, che diventa sostanzialmente strategico per andare a definire definire le necessità dell'agricoltore, dopo aver lavorato per mesi e mesi la propria terra e aver prodotto un prodotto sano e salubre, per vederlo alla fine almeno remunerato nei costi. C'è il tema del contrasto alla PSA, che non significa solo ed esclusivamente fauna selvatica, perché a volte, quando ci ritroviamo in Commissione o nell'interpretazione legislativa dei

combattere la peste suina africana e arrivare nei prossimi mesi ed anni all'eradicazione. L'altro tema sostanziale è mettere in sicurezza gli allevamenti attraverso un piano strategico nazionale sulla biosicurezza, foreste (Masaf), che darà delle risposte puntuali in questo settore. Vengo al tema della siccità. È vero che quest'anno in gran parte del Paese abbiamo problemi più alluvionali che non siccitosi, ma c'è una parte che ha problemi di siccità (l'anno scorso tutto il Paese aveva questo

il piano da 13 miliardi per i primi 950 milioni di euro. In questo provvedimento c'è un'identificazione puntuale per dar vita alle progettualità.

a delle pericolose vertenze con gli enti pubblici e, dall'altra parte, senza essere sotto scacco di una normativa che non è così chiara a livello nazionale. Oltre a questo, abbiamo previsto anche delle misure per quanto riguarda gli adempimenti assicurativi. C'è il tema della siccità e quello della cabina di regia per quanto riguarda la protezione del nostro Paese dalla carenza di acqua,

proprio in questi giorni per misure emergenziali alla Sicilia attraverso un emendamento importante - è fondamentale, così come far funzionare bene il Fondo Agricat e tutto il sistema assicurativo. Abbiamo un problema enorme e lo sappiamo tutti: le compagnie di assicurazione non vogliono più indennizzare l'agricoltura perché sono in forte perdita. Quindi, o andiamo a realizzare un sistema come questo, efficiente, puntuale, pubblico-privato insieme a sostegno dell'agricoltura, oppure non avremo modo di proteggere le produzioni agricole italiane. Sottolineo anche l'impegno dei commissari, che voglio ringraziare, sulle tecniche di evoluzione assistita, con la proroga di questa sperimentazione che auspico. Come ha detto prima il Presidente, non siamo andati troppo oltre la scadenza di cui all'emendamento, perché speriamo di dare un procedimento strutturale in modo che tutti i nostri produttori e i nostri coltivatori possano usufruirne.

onorevoli colleghi, unitamente alle altre forze politiche dell'opposizione e ai Gruppi di opposizione, abbiamo deciso di presentare la questione pregiudiziale su questo provvedimento per una serie di ragioni. Prima fra tutte,

di fatto legifera e il Parlamento deve solo discutere e ratificare quello che il Governo decide. Questo è il dato fondamentale: certamente c'è

Questo non riguarda solo il rapporto tra il Parlamento e il Governo, ma riguarda davvero i valori e i diritti fondamentali della Carta costituzionale, che assegna al Parlamento e agli eletti la priorità della discussione, non la ratifica: questo è il dato. C'è una differenza tra la costruzione della proposta, delle soluzioni e la decisione, come ho già detto altre volte, ovviamente tra la maggioranza e l'opposizione, però il problema è che ratificare significa ridurre il ruolo del parlamentare e del Parlamento. Noi assistiamo sistematicamente allo svilimento del Parlamento e delle sue funzioni nell'accentramento delle funzioni legislative nel Governo. In sostanza, state già

Passiamo ad evidenziare alcune forti criticità in relazione ad alcune specifiche disposizioni del decreto-legge: ad esempio, l'articolo 4, in tema di rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, in merito al quale è del tutto inopportuno il ricorso allo strumento d'urgenza, tanto più grave se si considera la mancata adozione già lo scorso anno - e anche quest'anno - della legge annuale sulla concorrenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, degli articoli 101 e 109 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 47 della legge 23 2009, n. 99. In sostanza, una legge che non applicate la fate diventare una decretazione d'urgenza. Questa è davvero una cosa che grida vendetta dal punto di vista del principio costituzionale. Inoltre, come ho già detto in altre occasioni, sono state introdotte numerose norme che rendono ancora più eterogeneo il contenuto del provvedimento, con svariati profili di delicatezza e complessità, che vanno a incidere direttamente, non solo nel merito, ma anche sulla tenuta dei principi costituzionali.

devono scegliere tra avere un posto di lavoro e, nello stesso tempo, magari morire per un tumore, oppure morire di fame perché non hanno più un posto di lavoro. Non spetta ai cittadini compiere questa scelta. I cittadini devono avere la possibilità di avere un lavoro sano in un ambiente sano. Questo vuol dire affrontare il problema di quale sia l'indirizzo strategico di questa impresa. Come si pensa di rilanciarla:

ovviamente, noi contestiamo questa impostazione in violazione anche di quello che voleva essere il decreto stesso. Poi vi sono gli articoli 9 e 10, riguardanti

disposizione che tante polemiche ha suscitato: i giornali li leggiamo tutti. Tant'è che era stato espunto dal testo prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, a riprova della totale

ma oggi non potete farlo. La Costituzione vigente in Italia è quella che non è ancora stata modificata. Quindi, il Parlamento è centrale dal punto di vista della discussione.

Grazie, Presidente.

Ieri abbiamo discusso e votato un decreto-legge sulle rappresentanze sindacali dei militari; un decreto-legge sull'agricoltura. Ora, gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono proprio molto chiari e stabiliscono che la funzione legislativa appartiene al Parlamento, ma queste sono proprio nozioni base di diritto costituzionale: il Governo dovrebbe fare l'esecutivo, il Parlamento dovrebbe fare il legislativo. piccola distinzione - ironizzo, signora Presidente - ce la siamo persa ormai da tempo e non possiamo farne soltanto una colpa a questo Governo, per carità, tant'è che in alcuni tentativi di riforma costituzionale del passato si è provato a risolvere il tema della iperdecretazione d'urgenza anche, per esempio, creando creando i disegni di legge a data fissa, in modo tale da poter mettere il Governo in condizione di portare avanti i provvedimenti chiave del proprio programma nella certezza della tempistica. Tutto ciò senza tirare per la giacca l'istituto della decretazione d'urgenza,

creato reati per decreto-legge, quindi reati che sono diventati tali, incidendo sullo statuto di libertà dei cittadini dopo un semplice Consiglio dei ministri, e che sono stati anche poi modificati in sede di conversione grazie a emendamenti del Governo stesso, che quindi ha ammesso di averli scritti male. modo, abbiamo avuto figure di reato che hanno vissuto nel nostro ordinamento perché il decreto-legge era già in vigore, ma nei sessanta giorni quella stessa figura di reato si era modificata, con problemi enormi per gli interpreti, per i giudici, di applicazione dei principi della successione delle norme penali nel tempo. Questo è successo, così come è successo, come abbiamo visto ieri, che si sia utilizzato lo strumento del decreto-legge per norme puramente ordinamentali. Signora Presidente, mi aiuti a capire per quale motivo si deve varare un decreto-legge per stabilire i distacchi dei militari che sono assegnati alle rappresentanze sindacali o la misurazione della rappresentatività di questa o di quella sigla sindacale, quando si tratta di norme che potevano essere quasi stabilite con una circolare ministeriale. Tra l'altro, trattandosi di provvedimenti pacificamente accolti, perché anche le opposizioni più dure si sono astenute e quelle più ragionevoli hanno votato a favore, quel provvedimento poteva essere preso tranquillamente con un disegno di legge ordinario, che forse si poteva approvare addirittura in sede deliberante. Si trattava,

secondo la Costituzione non ci sono. Questa è una norma estremamente eterogenea, per esempio, che è stata imbottita come un *sandwich* durante l'esame in Commissione. Quindi si sono surrettiziamente fatte salire sull'autobus di questo provvedimento di legge anche norme che non avevano davvero niente a che vedere, per esempio, con l'agricoltura. Andiamo ad approvare norme sull'Ilva e sulle imprese strategiche per coprire il pateracchio che il ministro Urso sta facendo con ogni tanto lo vediamo arrivare qui, ma la situazione di Ilva è sempre peggiore e stiamo andando direttamente, signora Presidente - diciamolo in questa sede - verso la chiusura di quell'impresa. Quella è un'impresa strategica che il Governo si troverà

Questo Governo ha eliminato il reddito di cittadinanza, ma stiamo creando una specie di reddito di cittadinanza per gli abitanti di Taranto e provincia, perché alla fine quello che si vuole fare fare sostanzialmente è tenere quelle persone in cassa integrazione per sempre, senza avere neanche l'acciaio che serve a un Paese trasformatore ed esportatore come l'Italia. Ci sono norme sulla siccità, ci sono norme sulle malattie degli animali, c'è qualsiasi tipo di norma in un provvedimento che è assolutamente eterogeneo, quindi privo di quei criteri di omogeneità che un decreto-legge dovrebbe avere, non ha nulla di urgente, perché questo provvedimento non va a incidere su una specifica situazione

per poter creare quelle eccezioni al principio che a legiferare sia il Parlamento e a esercitare il potere esecutivo sia il Governo e quindi la incostituzionalità di questo provvedimento è evidente. Voglio aggiungere un altro punto, perché poi sembra quasi che si utilizzi questa strada anche per far fronte alle inadempienze del Governo stesso, perché sappiamo che abbiamo un obbligo: ogni anno dovremmo approvare una legge sulla concorrenza, signora Presidente. Questa maggioranza il concetto di concorrenza ha proprio dei problemi di tipo freudiano, tanto che se lo sognano la notte; sappiamo quanto l'idea di mettere a gara delle concessioni sia una cosa che dà agli esponenti della maggioranza delle vere e proprie palpitazioni, li mette in una situazione di aritmia cardiaca. Non so chi di voi abbia avuto oggi occasione di andare da qualche parte a Roma, ma di taxi sostanzialmente non c'era ombra. Poi abbiamo la ministra Santanchè che quando arriva alla stazione Termini si scandalizza, ma qualcuno dovrebbe ricordarle che fa il Ministro *en passant*, ma anche in tal caso

in questo decreto-legge, quindi, avrebbero dovuto più correttamente essere oggetto di quella legge sulla concorrenza che non si è fatta né l'anno scorso, né quest'anno. E invece che cosa si fa? Si utilizza sempre questa specie di *omnibus*, questa specie di veicolo, di veicolo, nel quale alla fine si infila di tutto. Naturalmente sappiamo che il Ministro dell'agricoltura ha una sua autorevolezza intrinseca che gli consente di fare un po' il bello e il cattivo tempo, ma questo non ci esime, come opposizioni, di dire che siamo in presenza, con questo malloppo, di una palese violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione,

in realtà sarebbe stato molto più utile e giusto che ciò avvenisse all'interno della legge annuale sulla concorrenza. Come però già anticipato dai colleghi, siamo fermi al 2022, con la legge votata nel 2023. Manca ancora la legge annuale del 2023

Signora Presidente, non tornerò su quanto detto dai miei colleghi. È semplicemente visibile, come ha detto il senatore Scalfarotto, guardando il fascicolo e leggendo il testo che c'è stato consegnato e quello che oggi presentiamo in approvazione, che essi non sono nemmeno figli o parenti di quello che è il testo originario se non in alcune parti. Riconosciamo in alcune parti

Si è colta l'occasione in questa strozzatura della democrazia che si è voluta realizzare con questo decreto di urgenza per fare dei *blitz* in ordine ad alcune fattispecie che erano state espunte in sede di prima

le proposte e le esigenze di confronto rispetto a temi che non incidono su di noi, ma sulla vita di tante imprese, di tante famiglie, di tanti territori che oggi non vedono risposte sufficienti. È evidente che questo continuo ricorso alla decretazione e il continuo ricorso

ma il popolo perché ci ha eletto? Ci ha eletto per prendere delle carte, leggerle, nemmeno discuterle e passarle da un ramo all'altro del Parlamento o per entrare nel merito delle fattispecie? Io credo che noi dobbiamo entrare nel merito delle fattispecie e dobbiamo anche avere il coraggio di confrontarci su di esse. Vorrei concludere dicendo che siamo partiti da un decreto elettorale o decreto di propaganda,

in fase di conversione, è diventato un decreto veicolo, dove sono stati scaricati centinaia di emendamenti (credo siamo arrivati intorno a 1.000), per poi arrivare in fondo

che al Gruppo Partito Democratico possa essere imputato di non aver tenuto un comportamento costruttivo in Commissione e di essersi sottratto alle sue responsabilità quando siamo stati chiamati ad approvare norme che erano nell'interesse del Paese. *(Applausi)*. Penso al florovivaismo,

Voglio concludere dicendo anche che, quando si mortifica la democrazia, questo non riguarda solo i deputati e senatori di opposizione, ma anche quelli di maggioranza, che ne subiscono le conseguenze. *(Applausi)*. È sufficiente andare a vedere la mole dei ritiri di emendamenti presentati per dimostrare che, quando non si esercita il modello democratico e parlamentare, come prevede la nostra Costituzione, i diritti mortificati sono quelli dei cittadini e delle imprese, ma anche quelli di chi è stato eletto per rappresentarli.

Vede, Presidente, questo decreto-legge è di fatto una norma *omnibus*, come è già stato detto negli interventi precedenti. I cinque capi dell'articolato disciplinano materie molto diverse tra loro, che in parte non hanno niente da spartire con l'oggetto del decreto-legge stesso. Pur sussistendo la necessità di far fronte ad esigenze reali e urgenti del settore agricolo e degli allevamenti - e do atto che alcune delle decisioni prese in questo decreto

dicevo, questo provvedimento è inadatto ad essere affrontato con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbe invece, come hanno detto i colleghi prima, nuove regole meditate meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, quindi con il pieno coinvolgimento del Parlamento anche nella fase di elaborazione. Viviamo però nel momento in cui il Governo si assume il ruolo legislativo e anche qui lo fa. Io intendo però concentrarmi su un tema e cioè sul problema della peste suina africana, in particolare sullo scellerato mancato coinvolgimento, in questo decreto, dei cacciatori nelle misure adottate per affrontarlo. Forse non è ancora abbastanza chiaro, ma ci troviamo in una condizione emergenziale e non sono più consentiti ritardi, errori ed omissioni nella strategia di controllo. Quando qualche anno fa furono constatati i primi casi di peste suina in Europa (in Belgio e in Slovacchia), si presero provvedimenti drastici sopprimendo ogni individuo di specie suine domestiche e selvatiche in un raggio di 5 chilometri dal focolaio individuato e, se la malattia non veniva debellata, allargando il raggio d'azione di tali abbattimenti; e non ci furono altri casi in quei Paesi. Da noi invece le decisioni della politica sono state, come troppo spesso accade, da un lato lente e farraginose, e dall'altro cerchiobottiste. Così, quando gli episodi di ritrovamento di cinghiali infetti si sono fatti frequenti in diverse regioni italiane, una serie di Paesi ha bloccato le importazioni dei salumi *made in Italy.* Con questo decreto-legge si prova a fare un passo in avanti. Mi chiedo però perché si coinvolgano l'Esercito e la Protezione civile, che nulla sanno di animali selvatici, e non i cacciatori in maniera formale, che sono gli unici esperti certificati di fauna selvatica. I cacciatori sono persone formate per legge e informate per interesse. Essi pertanto, più di chiunque altro, sanno come evitare di diffondere la malattia, che si trasmette per contatto con gli animali infetti e con le carcasse, disinfestando ogni volta con attenzione le attrezzature, gli abiti, le scarpe e i veicoli. Allo stesso tempo, i cacciatori, frequentando quotidianamente per passione i luoghi in cui maggiormente si concentra la presenza dei cinghiali, possono fungere da sentinelle del territorio, segnalando alle autorità competenti la presenza di carcasse o di branchi in prossimità di allevamenti di suini. Faccio allora fatica a capire perché, in questo provvedimento, non si sia seguito l'esempio di alcuni piani regionali, compreso quello della Provincia autonoma di Bolzano (che a suo tempo ho contribuito personalmente a pensare e a realizzare), e le richieste che sopraggiungono da diverse categorie di persone interessate dal punto di vista economico o professionale, coinvolgendo fin da subito - ed è comunque già tardi - i cacciatori. Appare evidente che sulla decisione politica di escludere i cacciatori incide l'imperante mentalità e la conseguente battaglia di diverse associazioni ambientaliste ed animaliste contro la caccia. La conseguenza è che non viene affrontato adeguatamente il problema, in prospettiva più grave per la nostra produzione alimentare *made in Italy*, che tanto sta a cuore all'attuale signor Presidente, che alcune Regioni coinvolgono i cacciatori, ma se i soldi che costano Esercito e Protezione civile fossero dati alle associazioni dei cacciatori, si potrebbe essere certi che il monitoraggio e il prelievo sarebbero fatti bene, per tempo e con efficacia. Va ribadito poi, come per altre situazioni dove è stato richiesto l'intervento dell'Esercito in ambiti civili, un concetto di fondo: le donne e gli uomini in divisa sono formati e pagati per altri scopi ed a quelli dovrebbero dedicarsi. Servirebbe qui invece un dispositivo articolato che valorizzi le persone con esperienza nel rapporto tra natura e attività umane, che preveda interventi rapidi e sburocratizzati: barriere, controllo del territorio, riduzione dei cinghiali selvatici, più controlli sanitari negli allevamenti, fino al rilascio di un vero e proprio *green pass* sugli animali oggetto di controlli campione. È chiaro che alcuni di questi interventi possono incontrare resistenze da parte delle associazioni predette; evidentemente, come spesso accade in simili casi, anche qui il decisore politico preferisce tenersi buone queste associazioni per evitare polemiche e sperare che l'Esercito, la Protezione civile e lo stellone italico aiutino a far rientrare la situazione. Ma accadrà difficilmente questo ed il grave è che nel nostro Paese ci sono precedenti che fanno da monito, come la Xylella fastidiosa, dove, per non voler intervenire drasticamente fin da subito, ci si è trovati dopo e ci si trova ancora nella condizione di abbattere migliaia e migliaia di olivi in Puglia: un vero e proprio disastro ambientale, economico e paesaggistico. Al contrario, l'avvento del colpo di fuoco batterico in Alto Adige a partire dal 1999 ha potuto essere circoscritto grazie al decisivo e rapido intervento pubblico, che ha fatto abbattere e distruggere migliaia di arbusti ornamentali appartenenti alla famiglia delle rosacee e facilmente infettabili, oltre al relativo numero di alberi di melo colpiti all'inizio, salvando però in tal modo milioni di alberi di melo e le conseguenti produzioni agricole. Questo a dimostrazione che, se la politica fa il suo dovere, anche a costo di apparire impopolare, si prevengono i problemi, altrimenti no. In questo caso, probabilmente no. Infatti, signora Presidente, la sensazione è che qui non si stia facendo tutto quello che è necessario e i costi ambientali, sociali ed economici di oggi non saranno nulla rispetto a quelli che si andranno a pagare un domani per la questione della peste suina. Spero naturalmente di essere smentito dai fatti, ma il mancato coinvolgimento dei cacciatori e in generale l'approccio non rigoroso al problema non fanno presagire il meglio. Signora Presidente, mi permetta di associarmi ai ringraziamenti del collega Franceschelli, ai funzionari degli Uffici della Commissione, ma anche al sottosegretario La Pietra, al presidente De Carlo e al relatore Bergesio per l'attenzione che hanno posto in Commissione alle questioni e alle proposte che abbiamo portato avanti. Purtroppo, tale attenzione non si è trasformata in un recepimento, anche in principio, di alcune delle questioni che abbiamo posto. Anzi, purtroppo, ancora una volta constatiamo che i colleghi di maggioranza approveranno un decreto ricorrendo all'annunciato voto di fiducia che svilisce l'azione legislativa dei parlamentari *(Applausi)*, di coloro che sono stati chiamati dal popolo per rappresentare in quest'Aula la voce mai univoca, ma sempre legittima, dei cittadini. Costringere al pensiero unico non è democratico e non è utile né al Governo, né al Paese. Abbiamo oltre 200 menti, signora Presidente, in questo ramo del Parlamento che - mi permetta di dire - sono in grado di pensare, elaborare e decidere sugli effetti futuri delle proprie decisioni, 200 menti che purtroppo i voti di fiducia bloccano. un Parlamento costretto ad eseguire il volere e gli ordini del Governo: che grande spreco di risorse. Purtroppo, stiamo vivendo la prefazione di quello che i partiti di Governo vorrebbero fosse il nuovo capitolo della storia repubblicana, il premierato, un capitolo che non ci piace e al quale ci opporremo, utilizzando gli strumenti democratici a noi disponibili. Il decreto-legge che esaminiamo oggi mette assieme due tematiche completamente diverse fra di loro: agricoltura e imprese di interesse strategico, tematiche certamente meritevoli di dignità maggiore e approfondimenti specifici. Il comune denominatore che troviamo nel modo in cui sono trattati nel decreto questi temi (per dire la verità anche molti altri temi) è la drammatica mancanza di una visione del futuro. Manca una programmazione strategica capace di rassicurare imprenditori italiani e stranieri, lavoratori e quelle centinaia di migliaia di famiglie che da questi settori traggono sussistenza. Per l'agricoltura il decreto propone provvedimenti che sono essenzialmente mirati a mettere delle toppe alle voragini che si aprono sotto la tempesta delle emergenze e della mancanza di prevenzione e programmazione. Con questo provvedimento non si fa prevenzione, anzi si cerca di curare in maniera approssimativa, con poche risorse e interventi incapaci di risolvere alla radice i problemi reali e da codice rosso. Due esempi su tutto sono il granchio blu e la peste suina: problemi che stanno mettendo in ginocchio gli operatori del settore e sui quali il Governo propone toppe temporanee, pur sapendo che si apriranno falle ancora più profonde che bisognerebbe prevenire con misure mirate e chirurgiche, le stesse misure che servirebbero per combattere seriamente un'altra piaga: il caporalato. Signora Presidente, il caporalato si contrasta e si previene seguendo due strade, entrambe indispensabili e necessarie. La prima è quella dei controlli severi, rigidi e costanti, non mossi soltanto dall'emozione del momento o dall'attenzione che i *media* riservano al problema per un evento tragico, come quello del barbaro abbandono e della morte del giovane bracciante emigrato Satnam Singh: evento, ma piuttosto omicidio, che ha scosso ognuno di noi per la brutalità con cui si è consumato. I controlli sono parte integrante del sistema come forma di prevenzione: non come tentativo di cura; prevenzione di un male che troppo spesso si insinua nella sottocultura offensiva e putrida dello sfruttamento del lavoratore, ancora meglio se straniero, alimentando l'ingordigia logica del profitto personale che considera tasse, contributi previdenziali e persino le assicurazioni come pizzo di Stato. No, signora Presidente, non si tratta di pizzo di Stato. Si tratta di rispettare la legge e di rispettare i lavoratori e le loro famiglie. Come a sua conoscenza, signora Presidente, abbiamo gli strumenti normativi per garantire sistemi di controllo su tutto il territorio nazionale. Servono maggiori risorse e la volontà politica del Governo, che ha il dovere di attuare le leggi che garantiscono la totale sicurezza sul posto di lavoro e il rispetto dei diritti al lavoro, alla dignità e alla vita. È una questione di civiltà. La seconda strada da seguire, per contrastare il caporalato, è quella, purtroppo non percorsa dal Governo, di creare un terreno fertile per chi segue e rispetta la legge. Dobbiamo garantire che rispettare le regole sia conveniente, non solo per evitare le multe, ma anche perché così si creano i presupposti essenziali per aprire le strade a finanziamenti, a benefici fiscali, alla pianificazione del futuro attraverso prospettive di crescita che lo Stato e l'Europa devono garantire. Come diceva il giudice Paolo Borsellino, signora Presidente: è chiaro che quanto più le leggi vengono osservate, tanto più si ritiene che siano giuste. *(Applausi)*. Gli emendamenti che noi del Partito Democratico avevamo presentato in Commissione andavano in questa direzione, suggerendo di usare la digitalizzazione, capace di snellire le attività burocratiche, che ci sembra ancora scarsamente considerata, se non guardata con diffidenza, da chi teme che la trasparenza possa frenare l'economia. Noi sappiamo che non è così. È l'inverso, signora Presidente. Sono le acque torbide a essere il regno di chi pensa che il profitto personale valga più della vita e dei diritti dei lavoratori. Abbiamo chiesto alla maggioranza di adottare il nostro emendamento, che avrebbe inserito il possesso del documento unico di regolarità contributiva come strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione o dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo e finanziamento. Lo abbiamo chiesto per lanciare un messaggio chiaro agli imprenditori onesti: lo Stato è con voi. Lo Stato vi tutela. Lo Stato vi premia. Lo Stato vi affianca nella lotta alla concorrenza scorretta. scorretta. I partiti di maggioranza non ci hanno dato ascolto. Signora Presidente, l'agricoltura presidente è un settore che contribuisce al 3,8 per cento del PIL italiano e al 3,6 dell'occupazione nazionale e alla diffusione del *made in Italy* nel mondo. Pensavamo fosse logico che nel decreto agricoltura si affrontassero questioni e interventi strutturali, anche per utilizzare al meglio i vantaggi competitivi che l'Italia offre nelle sue diverse e magnifiche Regioni. Un esempio, del quale abbiamo discusso anche la scorsa settimana, è il settore florovivaistico; un altro è la valorizzazione degli ingredienti della dieta mediterranea. Entrambi i settori sono tipici delle Regioni del Mezzogiorno, grazie al calore del sole e alle qualità organolettiche di terreno. Potrebbero quindi rappresentare un volano di occupazione e sviluppo di aree per noi strategiche. Ma di strategia, in questo decreto, non c'è ombra, né una benché minima traccia, come del resto accade per la politica industriale. Questo decreto, infatti, parla di imprese a interesse strategico. Ebbene, è la stessa parola "strategico" che contiene in sé l'obbligo ad affrontare l'argomentare con visione futura, seguendo un ben più ampio piano di sviluppo, capace di delineare con nitidezza il destino del Paese. Avremmo voluto che questo decreto facesse finalmente chiarezza sulla politica industriale di questo Governo. Avremmo voluto confrontarci sulle linee guida. condividendole o magari scontrandoci. Almeno, signora Presidente, avremmo fatto chiarezza. Invece, siamo ancora qui a chiederci: ma qual è la politica industriale di questo Governo? Non lo sappiamo noi, non lo sanno gli imprenditori, non lo sanno i sindacati e le associazioni di categoria, non lo sanno i possibili investitori italiani e stranieri, non lo sanno i dipendenti delle aziende. Il vero problema è che lo stesso Governo a non sapere quale sia la sua politica industriale: e non lo sa perché questa politica non esiste. Signora Presidente, questo Governo continua ad operare solo dove c'è un'emergenza, senza riuscire a risolvere il problema. Ebbene un'emergenza è quella dell'Ilva di Taranto. Ad oggi l'Ilva ha solo un altoforno in funzione. Una sentenza della Corte europea di poco più una settimana fa richiede interventi significativi per prevenire danni ambientali e alla salute umana. Servirebbero quindi interventi urgenti, decisi, risolutivi, ma il Governo continua a proporre misure tampone emergenziali, continua ad essere in balia degli eventi e del mercato, come fa con tutte le questioni in materia di industria.

abbiamo perso un'altra buona occasione: sviluppo del settore agricolo, riconversione industriale, utilizzo di nuove tecnologie e trasparenza. Ci sarebbe stato tanto di cui parlare e su cui confrontarsi per contribuire a migliorare le regole di un gioco che non appartiene ai partiti, ad una maggioranza o una minoranza, ma al Paese intero di sistema, società e comunità. Purtroppo, anche questo provvedimento si risolve in uno spreco di risorse e di tempo; tempo che l'Italia e gli italiani non hanno, perché viviamo tempi difficili in cui il mercato globalizzato non ammette pause o indecisioni. Abbiamo doveri a cui non possiamo e non vogliamo sottrarci, ma dai quali questo Governo cerca di estrometterci, penalizzando solo il futuro del Paese e quello dei nostri giovani. Certo, il Governo sopravviverà al test della fiducia, come è avvenuto fino ad oggi; vincerà grazie alla forza dei numeri e all'utilizzo strumentale delle procedure parlamentari, ma sarà una vittoria di parte, non dell'Italia e non certo degli italiani. Noi continueremo a vigilare e a lottare.

la Cenerentola della nostra economia e anche dell'economia europea, ma grazie al Governo guidato da Giorgia Meloni l'agricoltura italiana riacquista giorno dopo giorno dignità in Italia, ma soprattutto in Europa. Debbo dire che mai come in questo momento

Granaio Italia. Dobbiamo far fronte ad un problema importante qual è quello del mercato dei cereali, che ha raggiunto livelli bassissimi, al di sotto dei costi di produzione, che deve fare i conti non con le difficoltà climatiche e ambientali che ogni giorno si pongono di fronte alle difficoltà che già gli agricoltori hanno, ma con le difficoltà

poi ci ritroviamo trasformati sulle nostre tavole; prodotti che non rispettano i crismi a cui gli agricoltori italiani, attraverso protocolli e disciplinari, sono giustamente costretti, perché producono bene, rispettando

che finora non erano stati affrontati in forma significativa e concreta, come la peste africana che ha colpito i suini, la brucellosi per quanto riguarda i bovini, gli ovini,

nel coltivare le specie che consentirà di far fronte a problematiche come la scarsità idrica, come l'utilizzo quantità di concimi minerali, come l'utilizzo se non l'eliminazione di alcuni principi attivi oggi utilizzati per coltivare alcune specie vegetali.

si definisce negli ultimi anni imprenditore, ma l'agricoltore è un uomo che deve fare i conti non solo con l'impresa, non solo con i costi, non solo con le difficoltà, non solo con i bilanci, ma anche con una componente su cui non può incidere, che è quella che dipende dal cielo, dal cielo, da una situazione climatica fortemente cambiata, che spazia da bombe d'acqua, da grandi periodi di piovosità a grandi periodi di siccità. Anche in questo senso il decreto, con l'articolo 11, ha messo mano ai problemi critici legati alla siccità, segno tangibile di attenzione alla problematica. Lo stesso si può dire per quanto riguarda le

debellato, è dovuto veramente ad una inconsistenza umana che rasenta l'omicidio. Ebbene, queste cose non debbono più accadere. Anche attraverso questo provvedimento avremo particolare attenzione affinché episodi tristi, tragici

a te, cosa dire per avvalorare il lavoro svolto? È importante aver affrontato sin da subito queste problematiche

che consente di avere sulle nostre tavole un prodotto sano, di grande qualità, buono, che è poi il *made in Italy* che ci caratterizza in tutto il mondo. Ebbene, Presidente, che dire per ringraziare quello che è poi comunque un primo approccio alle problematiche? È proprio il caso di dire che chi ben semina ben raccoglie. bene; il decreto-legge agricoltura presenta sicuramente i presupposti per avere un buon raccolto. Li avremo tutti perché abbiamo anche un Governo guidato da un Presidente come Giorgia Meloni e un Ministro sensibile ai problemi della nostra agricoltura.

per il lavoro svolto in Commissione i relatori e l'assistenza che vi è stata da parte dei funzionari. C'è un tema però che è emerso con molta chiarezza: questo provvedimento, che era una decretazione d'urgenza,

che, sulla questione dell'emergenza e della siccità in termini assoluti, e in particolare con riferimento al Mezzogiorno, alla Sicilia e alla Sardegna, con questo

Io sono convinto che tutte le persone nella Commissione e in quest'Aula danno una risposta negativa a tale domanda. Se c'è una decretazione d'urgenza e la risposta non è sufficiente, i casi sono due: o il tema non era urgente e, nel caso della siccità, lo è, o le risposte sono inadeguate. Ciò significa che si sta facendo semplicemente propaganda. E questo è tanto più grave perché il settore del quale stiamo parlando - come sa benissimo il Presidente della Commissione - è caratterizzato da elementi di soglie di irreversibilità. Ci sono delle soglie, superate le quali, si avvia la desertificazione. Ci sono delle soglie, superate le quali, in acqua ci sono delle specie che non sopravvivono. Ci sono soglie, superate le quali, certi terreni non vengono più coltivati e certi lavoratori abbandonano

in campagna elettorale, una propaganda per la quale tutte le difficoltà che abbiamo avuto nel settore dell'agricoltura e nel settore della pesca in Italia sono dovute soprattutto agli interventi della Commissione europea, che viene vista come una matrigna legislativa che impedisce ai tanti ai tanti lavoratori di poter realizzare le proprie aspettative. Ebbene, rispetto a questa propaganda, ciò che oggi c'è nel decreto è una collezione di misure totalmente inefficaci, inefficienti e insufficienti. Sulla siccità, per esempio, non ci sono misure strutturali, non ci sono misure di emergenza e non ci sono misure compensative. Oggi in Sicilia l'allarme che viene lanciato è di danni che stanno raggiungendo i 2 miliardi, semplicemente come danni complessivi. Noi avevamo presentato degli emendamenti che riguardavano la viticoltura, il tema della vendemmia verde e il tema di recuperare tutta una serie di colture che sono andate al macero; bisognerà risostituire quel tipo di terreni, perché il ciclo climatico li ha danneggiati. Ebbene, non c'è stata alcuna risposta positiva su questo da parte del Governo, forse perché davvero non era una semplice *gaffe* quella del Ministro dell'agricoltura, che vede come una fortuna la circostanza che la siccità non riguardi le zone del Mezzogiorno e della Sicilia. Ma in questo caso, oltre alla fortuna, c'è la sfortuna la sfortuna di avere un Ministro che non riconosce la gravità della situazione in Sicilia e non riconosce l'opportunità degli emendamenti che abbiamo presentato. Più in generale, sulla questione del settore agricolo, davvero si pensa che tutta la questione del prezzo minimo sia risolta da questo articolo? Il tema non è semplicemente avere una previsione di quelli che possono essere i costi attesi, peraltro in assenza di variabilità climatica e di variabilità di importazioni ed esportazioni. Si può costruire l'idea di un costo atteso, ma il tema è come si distribuisce la questione della rendita tra la distribuzione finale, che decide i prezzi giorno per giorno, e e chi svolge prima l'attività di produzione. Ma questo significa un intervento vero sulla concorrenza e anche sulla concorrenza sleale, che sono due concetti diversi. Intervenire sulla concorrenza significa definire misure di incentivi e di concorrenza che tengano conto dei mercati geografici rilevanti sotto il profilo *antitrust*, delle differenze regionali, delle differenze di costo, dei costi di trasporto, ma anche della circostanza che i mutamenti climatici, per esempio negli ortaggi, agiscono anche sul *time to market*, cioè sul tempo in cui la concorrenza agisce. Dobbiamo dare agli agricoltori innanzitutto una distribuzione di rendita tale per cui veramente la maggior parte della rendita vada non al proprietario della terra, ma a chi lavora dentro

che non è stato analizzato. Io non sono convinto che il tipo di contratto che viene proposto dia gli incentivi sufficienti. Ci saranno incentivi da parte di molte imprese nazionali a comportarsi esattamente come si comportavano le imprese straniere, cioè a delocalizzare. Questa è un'altra questione che incide sulla concorrenza sleale, è un sleale, è un tema urgente. Ma effettivamente la risposta - come hanno detto i colleghi - doveva venire da un altro tipo di intervento, un intervento di tipo industriale-agricolo, che guardi all'intera filiera, che dia degli incentivi di aggregazione, ma che agisca soprattutto sul piano della distribuzione. Un altro pezzo di emendamenti che non è stato tenuto in considerazione riguardava l'elemento della pesca, in particolare gli strumenti sulla demolizione delle diverse imbarcazioni per diverse tipologie di categorie. Noi proponevamo sostanzialmente che le risorse che vengono date a una certa area geografica restino comunque in quell'area geografica per la demolizione delle imbarcazioni, indipendentemente dalla capienza rispetto alle diverse categorie. Questo ci sembra ragionevole, perché significa ridistribuire le risorse nei territori e non semplicemente sulla base delle dimensioni delle imbarcazioni. Ci sono alcune zone come la Sicilia in cui le imbarcazioni più grandi non ci sono e sarebbe corretto che le risorse destinate alla demolizione di quelle imbarcazioni restassero sul territorio, anziché andare altrove. tale proposito non siamo stati ascoltati. Sul capolarato ha detto benissimo il collega Giacobbe: c'è un tema profondo di regole,

Però, guardate, se certe cose avvengono, è perché viene meno la considerazione umana e basilare della persona come meritevole di dignità. Soltanto il concetto di una persona come proprietà può permettere fatti del genere, e difficilmente avvengono per la follia di un singolo, che certamente c'è stata. La nostra domanda da legislatori responsabili è che cosa abbiamo fatto noi per favorire e far sì che singole follie possano produrre siffatti eventi? Questa è la domanda che ciascuno di noi nella propria coscienza deve porsi. Quando rappresentiamo il migrante come un soggetto non soltanto senza dimora, senza dignità umana, poi troviamo qualcuno che approfitta della sua follia per fare quello che è accaduto. *(Applausi)*. Su questo la risposta non può essere costruire un *database*, anche perché il *database* c'era già. c'era già. La risposta su questo non è costruire un *database*: la risposta è un insieme di politiche dettagliate quali quelle che noi abbiamo prospettato la settimana scorsa in una interrogazione Camusso. In conclusione, qui si è persa effettivamente un'occasione, ma temo soprattutto che non siano stati colti l'urgenza e il tema della irreversibilità. Vi parlo da siciliano: abbiamo tanti casi di desertificazione e qualche giorno fa abbiamo dichiarato morto il lago di Pergusa, raccontato da poeti greci e latini. Quello è un esempio di come la desertificazione avanza e non ci può essere cittadinanza quando c'è desertificazione; non ci può essere sovranità neanche alimentare quando c'è desertificazione. Mi auguro che, quando ci sarà il G7 a Siracusa, non si faccia vedere in Sicilia, ai nostri *partner* stranieri, ciò che in Sicilia anche da questo Governo non è stato fatto.

Nella conversione in legge di quel decreto-legge, grazie al senatore Luca De Carlo e con la quasi unanimità della Commissione agricoltura, fu aggiunto l'articolo 9-*bis* che semplifica le procedure per la sperimentazione in campo aperto di piante ottenute da nuove biotecnologie agrarie. Questa è stata una semplificazione importante che rispondeva a un'esigenza molto diffusa nella comunità scientifica di settore, molto sentita anche dagli imprenditori agricoli, visionaria, ed io stessa la salutai come una buona notizia. grazie a quella legge, il 13 maggio scorso si è inaugurata presso l'azienda agricola Radice Fossati a Mezzana Bigli, in provincia di Pavia, la sperimentazione in campo di una varietà di riso - è stata la prima volta - che potrebbe consentire di diminuire l'uso degli agrofarmaci; una sperimentazione messa a punto dalla professoressa Vittoria Brambilla dell'Università statale di Milano, tramite la tecnologia CRISPR-Cas9. È stato davvero un traguardo importantissimo per la nostra ricerca pubblica; un traguardo che si è realizzato in quella giornata che si è trasformata - eravamo presenti anche il senatore De Carlo e la sottoscritta - in una festa che, celebrava, oltre a quel traguardo importante, qualcosa di inedito nel nostro Paese e troppo poco frequentemente realizzato, e cioè un'alleanza tra scienza e politica. È la dimostrazione che, quando ci si allea, i risultati arrivano. Quella legge però aveva il grosso limite di imporre alle procedure semplificate per le biotecnologie in campo un termine, quello del 31 dicembre 2024, che la rendeva - io avevo usato queste parole - un'apertura mutilata. All'epoca presentai un emendamento per rendere permanente quella semplificazione, perché chiunque fa ricerca sa benissimo che un anno e mezzo non è sufficiente per valutare la resa delle condizioni e delle sperimentazioni in campo aperto di quelle culture e chiunque, anche non esperto in ambito agrario, può ben intuire che i cicli della natura non si conciliano con termini amministrativi puntuali, al 31 dicembre di qualsiasi anno. Questi erano già due elementi direi sufficienti da soli a far comprendere che sarebbero stati necessari nuovi interventi legislativi per non vanificare gli effetti di quella semplificazione e permettere, quindi, una programmazione delle attività di ricerca. Senza contare - come già citato - che già allora, a maggio del 2023, era in corso l'*iter* di una disciplina europea in materia di nuove biotecnologie vegetali, vegetali, che è in via di approvazione, e questa disciplina europea, entrando in vigore, andrà in ogni caso a sostituire quella italiana. Ebbene, un anno dopo il decreto-legge siccità ci ritroviamo di nuovo in quest'Aula chiamati a convertire un nuovo decreto in materia di agricoltura e i relatori in Commissione, i senatori De Carlo e Bergesio, meritoriamente hanno presentato un emendamento, che è stato approvato, per ampliare, da una parte, l'ambito delle possibili sperimentazioni e per prorogare di un altro anno, fino al 31 dicembre 2025, il termine alla semplificazione delle sperimentazioni in campo aperto di cui stiamo parlando. Io non posso che nuovamente felicitarmi con loro per l'interesse e il lavoro profuso su questa materia, tanto importante per la ricerca italiana e per l'ambiente, ma parimenti non posso che presentare lo stesso emendamento che presentai lo scorso anno per eliminare, anziché differire, questo limite temporale e rendere permanente la semplificazione delle procedure per poter far ricerca sulle biotecnologie nuove vegetali in campo aperto. Del resto, non ci sono argomenti scientifici per dover rendere nuovamente temporanea e non permanente una procedura che libera la possibilità di studiare la resa in campo aperto delle colture geneticamente migliorate; una libertà di ricerca che - lo ricordo - per più di vent'anni è stata ostacolata da un divieto di fatto. Ci sono studiosi, ci sono imprenditori in tutto il Paese che lavorano su vite, limone, frumento, pomodoro; su queste e altre culture tipiche italiane gli scienziati del nostro sistema hanno lavorato per anni e vorrebbero poterne valutare la resa con rigore scientifico, massima sicurezza e il tempo necessario per farlo. È chiaro che la posta in gioco è tutto: la conoscenza, lo sviluppo, la competitività del Paese, in un settore oggi vitale per mantenere la competitività della nostra In questo contesto è anche bene citare - l'ha fatto il senatore De Carlo - che venerdì 21 giugno l'Italia della scienza e dell'innovazione, ma anche la politica della scienza e dell'innovazione, si è svegliata con la pessima notizia che la coltivazione sperimentale della professoressa Brambilla era stata vandalizzata e devastata da ignoti ecoterroristi: una notizia che ha avuto risalto nel mondo dalle pagine della prestigiosa rivista «Science». Eliminare il limite temporale alle sperimentazioni in campo sarebbe vitale, sarebbe vitale, tanto più dopo questo atto vile, violento e oscurantista e sarebbe un segnale importante per la comunità scientifica italiana - a cui per tanti anni è stato impedito di condurre le proprie ricerche - del fatto che l'Italia è e vuole essere sempre di più un Paese che tiene nella giusta considerazione la scienza, la ricerca e i nostri studiosi. *(Applausi)*.

e nasconde sotto il tappeto i problemi veri. Penso sia giusto ricordare a tutti noi che i nuovi impianti ex Ilva sparsi nel territorio nazionale occupano direttamente più di diecimila lavoratori e coinvolgono non meno di ventimila tra indotto e altre attività. Tra questi ci sono quotidianamente, in cassa integrazione e smaltimento ferie, tra 3.500-4.000 lavoratori e lavoratrici. In capo all'Ilva ci sono poi 2.000 persone a cassa integrazione a zero ore. Riguardo all'indotto diretto, che coinvolge almeno 5.000 persone solo a Taranto, anche nell'indotto si fa ampio uso degli ammortizzatori sociali e in alcuni casi i lavoratori sono stati licenziati per chiusura dell'azienda per mancanza di commesse per crediti eccessivi che hanno messo in fallimento le aziende dell'indotto. Stiamo parlando sostanzialmente di oltre 30.000 persone e, quindi, di quante famiglie vengono coinvolte e cosa significa per l'Italia e il nostro Paese

servirebbe prendere una volta tanto in mano il problema dell'Ilva, fare una discussione pacata tra tutti noi, proprio perché ovviamente la situazione è a mio avviso - drammatica da questo punto di vista, e si corre il rischio di avere un'azienda di grande importanza che viene meno e il pericolo dal punto di vista della desertificazione industriale. È inutile dirlo: questo

Questa è la situazione che abbiamo se registriamo il disprezzo della vita umana, con il capitalismo razzista che c'è esplicita mettendo le persone nei casolari, nelle baracche, nelle tende e nelle roulotte. Facciamo finta tutti di non vederli. Questa situazione penso sia

Vorrei sottolineare a tutti noi che la scorsa legislatura era stata chiusa con una relazione di un'indagine conoscitiva sul caporalato che indicava molte cose da fare:

gli unici a pagare sono i lavoratori schiavizzati e sfruttati, ma anche gli stessi agricoltori, in particolare i piccoli agricoltori. Allora, forse, bisogna affrontare il problema in modo diverso

ha la soluzione in tasca. Non vi è, però, bisogno non di un decreto-legge, ma di una discussione seria su come è strutturata la filiera del prodotto in agricoltura, e non solo per poter dare una risposta

pretesa di avere la soluzione in tasca. Tutti noi in Parlamento, però, siamo chiamati a dare una risposta, perché da una parte ci sono 30.000 lavoratori e le loro famiglie che rischiano il posto di lavoro e, dall'altra, c'è un modo produttivo in cui il caporalato è diffuso e non solo nelle aree del Mezzogiorno, ma in tutto il Paese. Si tratta, quindi, di una piaga alla quale siamo chiamati a trovare una soluzione. iscritta a parlare la senatrice Licheri tenere sostanzialmente a galla lo stabilimento siderurgico ex Ilva. E io, Presidente, proprio sull'impianto tarantino ho concentrato il mio intervento, lasciando poi ai colleghi la trattazione del cuore del provvedimento. Intervengo sull'ex Ilva perché ritengo debba essere sfruttata ogni occasione per ribadire quanto inutile e inefficace si stia rivelando la politica industriale di questo Governo. Nello specifico su Taranto, è evidente che il Governo stia inseguendo gli eventi sul tema dell'ex Ilva. Tra Acciaierie d'Italia ed ex Ilva, la continua scelta di spingere per un finanziamento delle misure straordinarie non sta aiutando. Si continua a spostare in là la palla, evitando la discussione definitiva, ossia cosa fare del polo di Taranto. Servono tanti milioni - lo abbiamo detto e ridetto - per far tornare il polo Tarantino alla sua capacità ordinaria, ma il decreto ne stanzia soltanto 150; tutto questo dimenticando o forse, peggio, ignorando le problematiche ambientali e sanitarie. Di decreto in decreto, il Governo Meloni prosegue senza un credibile progetto di politica industriale e non chiarisce nulla sulle prospettive di tutela occupazionale, dei livelli di salute pubblica, di sviluppo economico, di tutela ambientale. Quali sono quindi le intenzioni? Qual è il progetto? Il Governo vuole rimettere l'acciaio al centro di un piano di strategia industriale? Non c'è chiarezza. Il destino dell'ex Ilva va assolutamente riscritto. È necessario lavorare affinché smetta di essere un caso emblematico negativo. Se ci pensate, ciò che racconta questo impianto ha del paradossale: ci sono state condanne, la magistratura ha disposto sequestri e ciò nonostante si è cercato in tutti i modi di mantenere in vita l'impianto a fronte, poi, di cosa? Di impegni improbabili, di promesse incerte.

residenti soffrono di livelli elevati di malattie respiratorie, malattie cardiache, cancro, malattie neurologiche debilitanti e mortalità prematura». E l'Italia invece cosa fa, tornando al paradossale di cui parlavo prima? Riconosce per legge l'immunità amministrativa e penale alle persone incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia ambientale. Si è cercato poi successivamente di ammorbidire in qualche modo i contenuti di queste previsioni con formulazioni

Ci troviamo nuovamente a discutere del suo futuro e l'orizzonte ad oggi è nero per l'occupazione, per l'economia, per il fronte ambientale, per quello della salute. La priorità, Presidente, è evitare quindi la chiusura di un impianto che contribuisce indirettamente all'1,5 per cento del PIL italiano? Ce lo chiediamo. Transizione energetica, difesa delle condizioni ambientali dell'impianto, lotta per un lavoro dignitoso e ben retribuito, strategia industriale seria per non ridurre le prospettive produttive e la quota di acciaio sfornata dagli altiforni: questi devono essere gli elementi che devono camminare e andare di pari passo e ogni capitale privato che vuole sostituirsi alla fallimentare gestione ArcelorMittal acciaierie d'Italia deve essere contenuto e perimetrato dallo Stato entro questi binari. Eppure, questo Governo non ha trovato niente di meglio da fare che tagliare gli investimenti. Sono stati bloccati 900 milioni per la transizione equa; ha cancellato un finanziamento di 1,2 miliardi di euro del PNRR necessari per la diversificazione industriale e ha letteralmente regalato 680 milioni di denaro pubblico ad ArcelorMittal prima di dichiarare lo stato di insolvenza. Ci chiediamo se è in questo modo che il Governo intende portare a termine gli impegni che si era dato. Così si va soltanto verso il baratro. Noi, Presidente, non vediamo altri scenari all'orizzonte. A farne le spese saranno ovviamente tutte le imprese dell'indotto che oggi sono a rischio chiusura. Ciò significa che più di 5.000 lavoratrici e lavoratori rischiano di rimanere a piedi mentre chi, tra loro, spera ancora di accedere alla cassa integrazione non ha alcuna certezza di tornare a lavoro, e intanto a Taranto le persone continuano ad ammalarsi; persone e cittadini che sono costretti ancora a scegliere tra lavoro e salute. All'amministrazione straordinaria era stato chiesto di predisporre e compilare un piano industriale, ma qui Signor Presidente, manca totalmente una strategia industriale nazionale. È come se ci fossero delle difficoltà e delle resistenze a capire e acquisire consapevolezza della necessità di un piano che tenga conto delle fonti inquinanti, delle bonifiche, della decarbonizzazione verso un progressivo abbandono del fossile per energie rinnovabili rinnovabili meno inquinanti. Una riconversione avrebbe ricadute positive non solo sul lavoro, ma anche e soprattutto sulla salute dei cittadini che oggi vivono a stretto contatto con polveri altamente inquinanti, dannose -come abbiamo detto e continueremo a dire - per la loro salute. Bisogna dirlo e basta. È stato già pagato un prezzo altissimo in termini di vite, soprattutto dei giovani. C'è un dato, Presidente, fornito da Legambiente che preoccupa molto: nell'anno appena trascorso la produzione a Taranto per la prima volta è scesa sotto i 3 milioni di tonnellate, però i livelli dell'inquinamento sono aumentati. Lo dimostra il fatto che livelli di PM10 e benzene nell'aria tarantina sono passati da una media annuale di 3,3 microgrammi per metro cubo di aria nel 2022

Il Governo Conte II aveva già intrapreso una strada per la riqualificazione del sito; una strada che questo Governo ha abbandonato, e non si capisce Il Governo Meloni è stato capace - dobbiamo dircelo - di farsi prendere in giro da ArcelorMittal che oggi investe in Francia, nella decarbonizzazione dell'acciaieria di Dunkerque, per una cifra di almeno un miliardo di euro, una beffa doppia se si considera che il Governo di Parigi ha promesso un investimento di 850 milioni di euro. Noi invece abbiamo regalato milioni di euro per farli andar via. Tutto questo continua ad essere paradossale. Che destino, che futuro ha la produzione nazionale dell'acciaio? Noi non siamo ostili a priori al mantenimento della produzione dell'acciaio. Quello che è però fondamentale e determinante è l'attenzione che deve essere data ai *dossier* industriali e ambientali. In quali condizioni verrà prodotto e quale futuro si vuole indicare indicare per l'Ilva? A preoccupare sono infatti le condizioni infrastrutturali degli impianti. Senza investimenti e senza manutenzione rischiano i tarantini e rischia l'intero Paese. Ricordo che l'ex Ilva di Taranto è tra le poche rimaste a ciclo integrale e, se vogliamo che sia competitiva sul mercato, non possiamo prescindere dall'avvio di un processo di decarbonizzazione. Sono gli stessi sindacati dei lavoratori che hanno sottolineato l'importanza di effettuare al più presto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Senza questi interventi a breve noi ci ritroveremo ad affrontare l'ennesima emergenza. Dobbiamo pertanto tornare a pensare e programmare un'agenda nazionale per le infrastrutture. In questo senso il PNRR è una grande opportunità perché impone piani e progetti di lungo corso; un'occasione che non possiamo perdere se vogliamo che il nostro Paese sia autosufficiente nell'industria dell'acciaio. Alle porte abbiamo la concorrenza indiana e quella cinese. Davanti a noi abbiamo però anche un futuro in cui i settori cruciali (costruzioni, aerospazio, automotive) possono ridare all'ex Ilva centralità e con lei un progresso e un ruolo di primo piano anche al Paese. In chiusura, Presidente, colleghi, vorrei tornare sull'immediato futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva e ovviamente di quelli dell'indotto. Si impone, a questo punto, un intervento serio e concreto. Le risorse stanziate sono poche. In fase emendativa si è aperta la possibilità di utilizzare altre risorse, che però non sono state quantificate; ma, se consideriamo le perdite che il sito produce ogni mese, le possibilità che a brevissimo si parli di una nuova emergenza occupazionale sono davvero molto concrete. si dice patriota; però, a questo punto, in quanto tale abbia questo scatto di orgoglio e programmi un futuro concreto e salubre per i lavoratori e le loro famiglie, che hanno pagato un prezzo altissimo, ai quali lavoratori e alle quali lavoratrici noi a questo punto dovremmo chiedere tutti i

il decreto-legge agricoltura che ci apprestiamo a votare è un provvedimento di fondamentale importanza per il futuro dell'agricoltura e della pesca italiane. Purtroppo, come tutti sappiamo, la nostra agricoltura sta vivendo un momento particolarmente complesso e pieno di difficoltà, a causa della crisi economica che ha colpito il settore primario. Proprio per questi motivi il decreto-legge mette in campo una serie di misure urgenti e nuovi strumenti che serviranno a rafforzare le filiere e a tutelare il lavoro e la produzione delle aziende agricole italiane. Il provvedimento offre risposte puntuali e soluzioni concrete sia da un punto di vista normativo, sia da un punto di vista economico, dimostrando ancora una volta come la difesa dell'agricoltura e del *made in Italy* sia un'assoluta priorità per il Governo e la maggioranza di centrodestra. Entrando nel dettaglio, il provvedimento interviene in molti ambiti e affronta di petto molte questioni sollevate dal mondo agricolo. Tra le tante misure contenute nel testo di legge, voglio partire da quella che probabilmente è la più importante, perché riguarda un'azienda agricola su tre. Mi riferisco alla moratoria sui debiti, prevista dall'articolo 1 per tutte quelle aziende che hanno registrato una diminuzione di fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente. Stiamo parlando, secondo i dati forniti dalle associazioni di categoria, di una potenziale platea di 150.000 imprese, che potranno beneficiare per un anno della sospensione del pagamento della parte capitale delle rate dei mutui. Una vera e propria boccata d'ossigeno per migliaia di imprese che quotidianamente devono affrontare l'aumento dei costi di produzione e dei tassi di interesse bancari. Altre misure importantissime da un punto di vista economico sono quelle a favore delle aziende colpite dalla moria dei kiwi, che potranno accedere alle risorse del fondo di solidarietà nazionale, i ristori per le aziende colpite dalla flavescenza dorata e gli interventi per sostenere le filiere in difficoltà. A tal proposito, mi preme ricordare le risorse del fondo filiere, che saranno destinate ai produttori di grano duro, e le risorse destinate alle imprese e ai consorzi della pesca, messi in ginocchio dalla crisi economica generata dal granchio blu. Proprio sull'emergenza del granchio blu il provvedimento introduce finalmente anche la nomina di un commissario straordinario, per fronteggiare una situazione che oggi è sempre più drammatica e che mette a rischio la sopravvivenza di oltre 2.000 imprese nel solo delta del Po. Un'altra questione fondamentale sulla quale interviene il testo di legge è quella del contrasto alle pratiche commerciali sleali, con l'introduzione di un meccanismo che garantirà pagamenti più rapidi a favore degli agricoltori danneggiati da queste pratiche. agricoltura interviene con decisione anche sull'annoso problema della fauna selvatica, con lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro di risarcimenti e l'uso dell'Esercito per contenere l'invasione di animali selvatici. Il nostro auspicio è che queste importanti misure di contrasto alla fauna selvatica vengano ora sostenute con piani regionali straordinari di contenimento, per ridurre il numero eccessivo di cinghiali che assediano campi, stalle e strade. Una vera e propria invasione che, oltre a devastare le colture, rappresenta un serio pericolo per gli ecosistemi e la sicurezza dei cittadini. Basti pensare che i danni provocati dalla fauna selvatica ammontano a 200 milioni di euro all'anno, oltre al rischio di diffusione della peste suina. Un'altra novità fondamentale introdotta da questo decreto-legge sulla quale esprimiamo la nostra massima soddisfazione è lo stop al fotovoltaico selvaggio a terra *(Applausi)*, con il divieto di installazione di nuovi impianti sui terreni agricoli; una norma sacrosanta e di assoluto buon senso che ferma, da un lato, il consumo indiscriminato di suolo agricolo e, dall'altro, la speculazione dei grandi fondi di investimento che mettono a rischio la produzione agricola e la sicurezza alimentare del nostro Paese. nostro Paese. Sacrosanti sono anche gli emendamenti che introducono misure sempre più dure e più stringenti contro il caporalato, che rappresenta una piaga inaccettabile *(Applausi)* che va combattuta ed estirpata dal nostro Paese in maniera definitiva. definitiva. Fatti come quelli di Latina non si devono vedere mai più nel nostro Paese. Gentili colleghi, come detto in apertura del mio intervento, il decreto agricoltura ha il grande merito di intervenire in maniera efficace su molte questioni e di fornire soluzioni concrete a molti problemi. E lo fa all'insegna di una strategia d'azione che garantisce più risorse economiche, meno burocrazia e più regole certe a difesa dei nostri agricoltori. Una strategia che ci trova perfettamente d'accordo, perché finalmente viene data priorità alla sostenibilità economica delle aziende agricole. agricole. Se vogliamo dare un futuro all'agricoltura italiana, la prima vera questione da affrontare è quella della produttività e della redditività delle imprese. Basta, basta con le follie *green* tanto care alla sinistra italiana *(Applausi)* e ai burocrati europei. Basta con la falsa ideologia *green* che sta mettendo in ginocchio migliaia di aziende. La sostenibilità ambientale non si realizzerà mai se prima non viene tutelata è garantita la sostenibilità economica e sociale delle nostre imprese, dei nostri lavoratori e delle nostre famiglie. Aiutare chi lavora e chi produce, tagliare la burocrazia, abbassare le tasse, difendere con ogni mezzo il *made in Italy* e l'agricoltura italiana: questa è la nostra missione, queste sono le priorità politiche della Lega, queste sono le cose che stiamo facendo al Governo e che dobbiamo continuare a fare ogni giorno di più per costruire un'Italia più forte, più giusta, più competitiva, con buona pace delle chiacchiere inutili della sinistra. Signora Presidente, colleghi e colleghi, signor rappresentante del Governo, anche in questo decreto-legge prevalentemente dedicato ai temi dell'agricoltura avete voluto metterci - diciamo così - una spruzzata sull'ex Ilva. Ancora una volta un modo estemporaneo e inadeguato di affrontare quella che forse è la madre di tutte le crisi industriali di questo Paese e che, al contrario di quello che state facendo, avrebbe bisogno di un approccio organico e di respiro,

Un approccio organico che vi abbiamo proposto nel corso degli ultimi venti mesi, senza purtroppo trovare ascolto. Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti: Acciaierie d'Italia, dopo aver assorbito ingenti risorse pubbliche negli ultimi mesi, è oggi in amministrazione straordinaria. La produzione è in costante calo, così come gli ordinativi. Soltanto un altoforno è in funzione, mentre altri due sono stati fermati per ragioni di sicurezza e per mancanza di pezzi di ricambio. Crescono i lavoratori in cassa integrazione, non c'è liquidità per pagare le fatture di fornitura e i servizi per l'indotto. Insomma, un disastro annunciato che necessitava di un cambio di gestione immediato, venti mesi fa, e di investimenti da parte di un vero e proprio socio industriale interessato a rilanciare il sito e a risanarlo, innanzitutto dal punto di vista ambientale; ipotesi, questa, sempre rifiutata dal Governo in carica, che ha creduto alle promesse del *management* di Arcelor Mittal, ha ceduto alle loro richieste, ha sottoscritto un *memorandum*, salvo accorgersi, al momento della necessaria ricapitalizzazione di Acciaierie d'Italia, che in realtà non vi era nessuna intenzione di investire e di ricapitalizzare l'azienda. colleghi, è bene fare fino in fondo un'operazione di verità. Sì, perché forse abbiamo superato il limite per la sopravvivenza dell'ex Ilva; sì, perché le prospettive per il futuro sono assai deboli. La situazione di Acciaierie - non vi è dubbio - è oggettivamente drammatica e la scelta dell'amministrazione ed è stata densa di incognite. L'amministrazione fin da subito si è trovata a navigare in acque agitate e dall'incerto approdo e questa operazione di verità è tanto più necessaria anche oggi, alla luce di notizie riguardanti indagini in corso della Guardia di finanza. si aggiunge adesso la sentenza della Corte di giustizia europea, sulla quale ritornerò più avanti, ma che da subito evidenzia quanta discrasia vi sia tra i tempi della realtà e quelli del Governo, dove persino lo strumento del decreto-legge appare lento ed inefficace. Su questa vertenza si gioca la capacità del nostro Paese di definirsi ancora competitivo e di definirsi un Paese industriale. Ve l'avevamo detto in occasione della conversione dell'ultimo decreto che andava aperta una nuova fase per evitare il ripetersi degli errori compiuti nell'ultimo anno e mezzo. Noi vi abbiamo sempre offerto, per la verità, la disponibilità al confronto sul merito delle questioni, che purtroppo avete sempre eluso, non facendo tanto un torto a noi, ma un torto a Taranto, alla città, ai suoi cittadini, ai lavoratori e all'intero Paese. Avevamo detto che il piano industriale era indispensabile per comprendere e valutare aspetti decisivi sul futuro dell'impianto, perché parliamo dello stabilimento più grande d'Europa e di un settore produttivo fondamentale per la nostra economia, indispensabile per il funzionamento di altri settori manifatturieri e cruciale per l'occupazione. Così tornate invece sulla materia, dopo che vi avevamo detto questo, con un pannicello caldo, con qualcosa che non è una terapia, ma è una dilazione, una presa di tempo, quando di tempo non ce n'è più e, anzi, rischiamo di essere fuori tempo massimo. Ve l'hanno detto i sindacati ieri, non non tanto tempo fa: ieri, in un incontro al Ministero del lavoro hanno giustamente giudicato irricevibile la richiesta di cassa integrazione al buio per oltre 5.000 addetti, di cui 4.400 solo a Taranto. Vi è la legittima richiesta che prima vi sia la presentazione di un piano industriale, che non può essere subordinato all'accettazione di questi numeri di cassa integrazione.

ci sia il via libera al prestito ponte e che si affrontino tutte le questioni strutturali legate alla ripartenza. In Commissione industria ve l'avevamo proposto con i nostri emendamenti, che avevano appunto l'obiettivo di fornire qualche certezza. Abbiamo per esempio proposto - l'avevamo fatto anche nei precedenti decreti - di istituire presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo istituzionale con il compito di individuare e valutare i soggetti presenti sul mercato, eventualmente interessati ad acquistare gli impianti ex Ilva e ad investire in essi, attenendosi a determinati criteri, a partire da quello del rilancio occupazionale e industriale e soprattutto della tutela ambientale e sanitaria. fatto riferimento prima. Questo è ancora è più necessario, alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea. Anzi, alla luce di quella sentenza, questo tavolo sarebbe ancora più strategico quale strumento di raccordo tra le istituzioni, le realtà territoriali e le organizzazioni sindacali. Avevamo presentato una serie di proposte in merito alle garanzie della continuità produttiva, al mantenimento dei livelli occupazionali, sulla prosecuzione dei processi di decarbonizzazione e di bonifica, per i quali si rende necessario il pieno utilizzo di tutte le risorse che originariamente sono state destinate, sulla cassa integrazione, sulla salvaguardia dell'indotto, sulla valutazione dell'impatto sanitario ambientale e degli interventi posti in essere. Concludo, signor Presidente, ma su questo voglio soffermarmi ancora una volta. Se ci aveste dato ascolto nei mesi precedenti, quando in più occasioni abbiamo presentato questa proposta emendativa, probabilmente adesso non ci troveremmo nella difficoltà nella quale siamo rispetto alla sentenza della Corte di giustizia europea. Quella sentenza, infatti, ha stabilito che che la valutazione del danno sanitario deve fare parte integrante ed essenziale del procedimento di autorizzazione alla protezione e all'esercizio della stessa installazione; che l'emissione di sostanze nocive deve essere sempre considerata preventivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio; che di fronte ad una situazione di accertato pericolo, grave per l'integrità dell'ambiente e della salute, l'attività industriale deve essere sospesa. Ora la parola passa al tribunale di Milano, come sappiamo. Ma sappiamo anche che la strada è tracciata. Il Governo avrebbe dovuto darci ascolto per affrontare finalmente questa questione, accogliendo le proposte emendative. Così non è avvenuto e su questo decreto-legge verrà posta l'ennesima questione La vostra inadeguatezza, però, ci preoccupa sempre di più. Per questo, vi chiediamo di fare presto e di non giocare con la vita dei lavoratori, di Taranto e dei cittadini di quella città. Signor Presidente, ministro Lollobrigida, sottosegretario La Pietra, per me è un piacere e un dovere, da Capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione agricoltura, intervenire su un decreto-legge molto atteso e fortemente voluto, che racchiude alcune misure di fondamentale importanza per un settore vitale della nostra economia, simbolo delle nostre tradizioni, delle nostre radici, della nostra storia. Un settore fondamentale, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista identitario. Il decreto agricoltura, come è stato brillantemente evidenziato dal presidente De Carlo e dal vice presidente Bergesio, i due bravissimi relatori di questo decreto-legge contiene stanziamenti complessivi per oltre 350 milioni di euro, soltanto per il settore agricolo. Non va inteso come un sostegno economico *una tantum*, fondamentale all'interno di un quadro congiunturale particolarmente delicato, quale quello che stiamo vivendo, ma come un vero e proprio cambio di paradigma, coerente con la strada tracciata da questo Governo e dal ministro Lollobrigida da quando è iniziato questo percorso. Basti pensare, dal punto di vista economico-finanziario, ai 170 milioni di euro destinati agli aiuti alle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura, colpite dalla crisi di mercato indotta da eventi geopolitici. Basti pensare ai venti milioni di euro stanziati per contrastare la peste suina africana. Basti pensare ai dieci milioni di euro di stanziamento aggiuntivo destinati al fondo per la sovranità alimentare del 2025, anche per il 2026. Basti pensare ai 40 milioni di euro milioni di euro per la ZES unica per il Mezzogiorno per le imprese agricole come credito d'imposta. Basti pensare ai venti milioni di euro incrementati per il fondo per la qualità e la competitività della produzione dell'intero comparto cerealicolo. Basti pensare agli stanziamenti altrettanto significativi per contrastare la Xylella, la brucellosi ed altre assolute emergenze del comparto agricolo. in assoluta coerenza con il cambio di paradigma a cui facevo riferimento prima, sono da cogliere con grandissima soddisfazione le misure previste all'articolo 5, laddove vengono limitate le procedure di utilizzo del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra.

preferito i parchi fotovoltaici ai campi coltivati, che addirittura talvolta hanno sovvenzionato gli agricoltori pur di non coltivare e di consumare il suolo, nella logica

il tema del contrasto alle pratiche commerciali sleali, con l'introduzione del costo medio di produzione previsto dall'articolo 4, per evitare le dinamiche, a volte davvero folli, della formazione del prezzo del prodotto e del suo lievitare da pochi centesimi di euro al chilo fino a 5, 6, 7 euro soprattutto sui banchi della grande distribuzione. Il collega Salemi sa meglio di altri quello che puntualmente è accaduto, soprattutto all'interno di alcuni contesti temporali per alcuni prodotti di eccellenza (penso al pomodorino di Pachino), laddove quello che ho prima esternato si verifica puntualmente. Per questo credo che sia molto importante, anche su questo tema,

del controllo di queste procedure, con un potenziamento radicale, sancito attraverso alcuni ruoli importanti attribuiti ai direttori di mercati generali, che dovranno segnalare la mancata trasparenza delle contrattazioni all'ispettorato centrale della tutela della è quanto previsto dall'articolo 1, attraverso il quale si determina la moratoria di dodici mesi sui mutui, includendo anche i prestiti e le cambiali agrarie, nel caso in cui le imprese agricole e della pesca abbiano subito perdite di volumi d'affari di almeno il 20 per cento In questo caso, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, viene riservato un contributo in conto interessi di 20 milioni di euro nel 2024, di 10 milioni nel 2025 e di 10 milioni nel 2020. Da siciliano, signor ministro Lollobrigida, non posso che apprezzare l'intervento previsto sul tema della siccità. In Sicilia è un'assoluta emergenza, caro sottosegretario La Pietra, con conseguenze devastanti all'interno di tutto il comparto agricolo. Vi sono alcune fotografie nitide dell'esistente che certificano come il 70 per cento degli agricoltori abbia subito perdite significative, registrando una diminuzione del 45 per cento della produzione di mais e foraggi, del 30 per cento della produzione di grano, del 20 per cento per quella degli ortaggi, senza dimenticare le gravissime difficoltà degli allevatori. Per questa ragione non posso che accogliere con grande favore l'approvazione di un emendamento che è stato proposto dal sottoscritto, dal capogruppo Malan, dai colleghi siciliani Sallemi, Russo e Bucalo, volto a determinare un contributo significativo alle imprese agricole siciliane che, a seguito della siccità, hanno subito danni e non sono state coperte da assicurazioni. Esse potranno accedere a un fondo da 15 milioni di euro di risarcimenti che credo rappresenti ossigeno vitale all'interno di un quadro congiunturale particolarmente delicato. cento del territorio è a rischio desertificazione. Circa 850.000 persone, ovvero un quinto della popolazione siciliana,

c'è l'assoluta necessita, però, di un'azione coordinata fra il Governo nazionale e il Governo regionale, che si sta puntualmente avviando in Sicilia a seguito della dichiarazione emergenza, laddove sono stati stanziati i primi 20 milioni di euro e all'interno di questo decreto-legge si registra un rafforzamento del ruolo del Commissario per la siccità e soprattutto l'ampliamento dei suoi poteri per l'efficientamento idrico. C'è anche la necessità, però, di una visione su questo tema, che non può non può limitarsi ad affrontare l'emergenza, ma deve contribuire a risolvere il problema in maniera strutturale. Penso alla costruzione di dissalatori, come si sta facendo in Sicilia, Sicilia, penso al potenziamento della rete idrica e penso anche alla sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza a fronte di una risorsa assolutamente vitale. In Sicilia vi è una perdita all'interno della nostra rete del 51 I nostri invasi sono riempiti per una percentuale del 25 per cento rispetto al totale. Ecco perché credo che ci sia la necessità di un'assoluta sinergia che si sta puntualmente registrando fra il Governo nazionale e il Governo regionale. Altrettanto importanti - mi avvio alla conclusione, presidente La Russa - sono gli articoli aggiuntivi grazie agli emendamenti dei relatori sul tema del lavoro agricolo, del contrasto al fenomeno del caporalato; una risposta immediata che viene anche da alcuni episodi che che hanno molto colpito la pubblica opinione, anche con un rafforzamento dell'organico, con molte assunzioni immaginate e da qui a breve realizzate. Per tali ragioni, complessivamente non posso che esprimere un sentimento di sincera gratitudine nei confronti del Governo per quello che ha fatto e voglio complimentarmi con il presidente De Carlo, con il vice presidente Bergesio e con tutti i componenti della 9a Commissione per il lavoro svolto, che credo abbia contribuito a migliorare questo testo.

bloccare il fotovoltaico a terra, sostenere le imprese sui mutui, intervenire in tante situazioni di crisi e anche il prestito stesso dell'Ilva non fossero

le idee paghino e lo facciano anche quando le idee sono buone da parte dell'opposizione e quando sono condivise. Questa maggioranza e questo Governo non hanno non hanno sicuramente fatto a meno di rendere partecipi tutti della bontà delle idee. Penso, ad esempio, a Granaio Italia; anche

di sottoscriverlo se non ne avessero ravvisato l'urgenza. Il collega Spagnolli ci ricorda che altre Nazioni sono intervenute in maniera più precisa e più puntuale. Ricordo, anche sommessamente, che ci sono Nazioni dove si fanno anche meno controlli rispetto a noi e quindi risultano meno casi perché si fanno meno controlli. Non credo che in Francia non abbiano il problema della PSA, semmai, forse, non posso dirlo con assoluta certezza, fanno qualche controllo in meno di quello che fanno i nostri servizi veterinari che comunque lo fanno per la tutela e la salute non solo degli animali, ma anche degli uomini. Giacobbe ha affermato che manca una visione sul futuro. Può darsi che manchi anche una visione sul futuro. Mi dispiace che non ci sia, però se la visione che manca sul futuro ha consentito a questo Governo in due anni di stanziare le risorse che nessun altro Governo aveva previsto negli anni precedenti, non credo manchi la visione e sicuramente non manca la volontà di intervenire su quelle che lui definisce toppe e voragini, come quella del granchio blu e della peste suina, che forse ragionevolmente potevano essere contrastate - la prima sicuramente - se ci fosse stato un sistema di monitoraggio già presente, che invece non esiste. I colleghi della Commissione sanno che abbiamo attivato un'indagine conoscitiva per renderci conto se abbiamo sistemi di monitoraggio e soprattutto strumenti per poi intervenire. Il collega Nicita ha parlato di interventi insufficienti sulla siccità. Se ci fosse, ma credo che i colleghi glielo possano riportare, che è vero che questo non è un decreto-legge che interviene solo sulla siccità. Il collega Pogliese ha prima ricordato che l'emendamento a prima firma Malan, sottoscritto da tutti i nostri senatori siciliani, rappresenti comunque uno stanziamento di 15 milioni, che qualcuno potrebbe definire toppa, ma che qualcuno definisce forse buoni come l'acqua. Ricordo a tutti e soprattutto a me stesso che questo è il primo Governo che ha istituito un anno fa la cabina di regia sulla siccità. Non credo che la siccità sia un fenomeno scoppiato con l'avvento del Governo Meloni, anzi è qualcosa che si trascina da anni, che nessuno aveva mai pensato di risolvere in maniera strutturale. *(Applausi)*. Anche in tal caso però sono i fatti che smentiscono certe affermazioni e non Luca De Carlo.

sociali. È attento a quello che è lo sfruttamento delle persone soprattutto straniere in certi contesti. È un Governo che deplora anche l'utilizzo strumentale di certe cooperative degli extracomunitari e degli stranieri, come abbiamo avuto modo di vedere

precisa spiegazione circa la questione delle TEA, posso dire che anch'io, come lei ben sa, sarei iperpropenso ad avere una normativa che non abbia un limite temporale. La nostra è stata una proroga di un decreto siccità che l'anno scorso ci ha consentito comunque la prima sperimentazione a terra proprio nell'attesa di quello che diceva lei e, cioè, che l'Europa possa normare in maniera moderna un tema che ci consentirà e ci consentirebbe già adesso di affrontare certe tematiche, come quelle della siccità, che mettono fortemente in difficoltà questa Nazione, ma non solo.

di quello che era entrato. Certo, questo è il fratello maggiore. Maggiori sono sicuramente le risorse che, grazie al lavoro dei commissari, hanno arricchito il provvedimento che oggi, grazie a Dio e agli uomini, conta quasi mezzo miliardo.

verificato l'opportunità di inserire anche degli emendamenti a tutela della filiera dei fornitori, ma è sempre più complicato e sempre più difficile. Infatti una strategia comune ci porterà sicuramente ad avere una soluzione adeguata, penso nei prossimi mesi, perché questa produzione va difesa. È un interesse nazionale e questa Assemblea ha delle grandi responsabilità su questo, a prescindere dal colore politico. Un altro tema che, a mio avviso, è molto importante

di responsabilizzare le assicurazioni, perché emettano queste polizze e diano un sostegno all'agricoltura è estremamente importante e lei lo sa bene. Da sole le compagnie assicurative non possono più lavorare in agricoltura, perché hanno delle fortissime perdite. Occorre sostenere e aiutare l'intervento delle polizze da parte di chi aderisce a questo sistema e, dall'altra parte, avremo la possibilità di avere una garanzia sulla mancata produzione in agricoltura. Prima alcuni senatori hanno riferito che non riusciremo a definire un prezzo minimo. Ma non è un prezzo minimo, è il costo di produzione, che è tutta un'altra cosa. Anch'io all'inizio avevo intuito che dal provvedimento venisse fuori un prezzo minimo, ma, dall'analisi che

la possibilità di avere una garanzia sulle sue produzioni e sul prezzo di vendita, collegato finalmente al sistema. Avere la possibilità di formalizzare i contratti per i mercati diventa fondamentale, perché molte volte l'agricoltore parte, parte, va al mercato e non sa che prezzo avrà del prodotto finale. Un costo di produzione, abbinato a un prezzo finale certo, con un contratto vero: questo dà la possibilità di dare delle risposte concrete. Perciò anch'io sono soddisfatto di questo provvedimento e credo che avremo sicuramente la possibilità di vederne gli effetti nei prossimi mesi, anche perché - l'abbiamo detto in precedenza - con 600 milioni di euro spalmati in tre anni, 150 in Ilva e il resto in agricoltura, credo che sia stato fatto uno sforzo notevole

innanzitutto rivolgo un saluto e un ringraziamento a tutti i colleghi del Senato per il lavoro svolto anche nella fase preliminare alla redazione del decreto-legge, cioè nella fase nella quale, in un rapporto normale con il Governo, arrivano da tutti i banchi del Parlamento, sia in Aula che in altre sedi, consigli su come poter intervenire e migliorare i nostri settori di carattere strategico. L'obiettivo che ci diamo è esattamente il contrario di quello che da alcuni veniva sottolineato come un difetto di questo provvedimento: la mancanza di strategia. In realtà, questo Governo ha una visione e una strategia di fondo che

sociale e delle relazioni anche di carattere internazionale), dando all'Italia la possibilità di svolgere quel ruolo che, a nostro avviso, nel tempo la storia le ha assegnato, ossia contribuire attivamente allo sviluppo di un pianeta che abbia dei connotati che corrispondono a qualità della vita e benessere. Molti di questi argomenti fanno riferimento al nostro modello di vita, alla storia millenaria che appartiene al nostro popolo; una storia che è stata contaminata da tutte le culture che nel tempo hanno attraversato il nostro piccolo lembo di terra e che hanno lasciato a noi in eredità una forza, una capacità e una qualità che è invidiata da tutto il resto del mondo e che noi con generosità dobbiamo continuare ad offrire al mondo per quanto possiamo e sappiamo fare in ogni ambito, da quello della ricerca a quello della nostra cultura di produzione agroalimentare e di trasformazione, che credo siano oggettivamente considerate una eccellenza, non tanto e non solo da noi italiani ma da tutti coloro che chiedono di comprare italiano e di imparare da noi come si possano produrre cose così qualitativamente importanti e anche come controllare la sicurezza degli alimenti.

Commissione ha lavorato per migliorare un intervento di carattere normativo che ovviamente nella fase di decretazione richiede l'intervento successivo del Parlamento non solo per l'approvazione

con riferimento preciso allo scopo di una decretazione in via d'urgenza che è quello di andare ad affrontare delle emergenze. Alcune di esse sono emerse negli ultimi mesi ed altre mesi ed altre in realtà, pur essendo presenti nell'attività d'impresa o nella vita sociale, erano state probabilmente affrontate con strumenti inidonei a risolvere i problemi. Non è detto che

pragmaticamente affronta alcune contingenze e mette alcuni punti fermi su alcune situazioni inevase che andrò a descrivere che potrebbero essere delle soluzioni. Se non lo saranno, andremo ancora ad intervenire perché lo siano, senza rinviare il problema ad altre legislature, come evidentemente è avvenuto in passato. Voglio ringraziare il sottosegretario La Pietra, che ha presenziato ai lavori della Commissione, e il collega ministro Ciriani *(Applausi)*, che hanno avuto anche una relazione istituzionale con tutti i luoghi delle decisioni rispetto all'azione che che la politica può svolgere, secondo un mandato che la Costituzione ci assegna per quota parte e che deve rispettare, nel complesso, quelle precauzioni che, rispetto a un provvedimento di questa natura, non devono mai trasformare un mezzo in un modo per aggirare altri modi di legiferare che sono insiti nella natura normativa che è assegnata prioritariamente al Parlamento e solo in via d'urgenza ad altri strumenti, che, come questo, accelerano le modalità

chiunque sia in grado di dimostrare che c'è stato negli ultimi trent'anni un Governo che in venti mesi ha messo più risorse sull'agricoltura di quanto ha fatto il Governo Meloni ce lo dica, ce lo dimostri e noi saremo ben lieti di dire che ci siamo sbagliati. Ma a noi risulta che questo Governo è quello che ha rimesso al centro l'agricoltura in Italia, con stanziamenti mai visti da alcun Governo degli ultimi trent'anni, o almeno da quando faccio attività politica, senza dovermi rivolgere alla storia della Nazione. Penso che possano bastare per ricordare alle forze politiche presenti quanto sia importante far seguire a delle enunciazioni delle questioni di carattere concreto: una di queste è lo stanziamento finanziario. Credo che sia oggettivo che di agricoltura, durante questi venti mesi scarsi di Governo, si sia parlato molto di più che nel passato, non solo perché sono emerse alcune problematiche e criticità di carattere generale, ma perché le scelte di questo Governo sono state orientate a capovolgere quella che era la visione di un'agricoltura che non avesse più il ruolo che gli è stato assegnato dalla storia e da chi aveva contezza del ruolo degli agricoltori. Parlo anche del livello europeo: un'Europa che nasce da trattati molto rilevanti e importanti, non tanto per la scelta di verticalizzare e rendere politico un contesto geografico, ma perché si davano degli obiettivi per rendere più prospera la vita dei cittadini. Faccio riferimento al Trattato di Roma in particolare, che nascono, sempre in Italia, con le linee guida di Messina. Le normative sull'agricoltura vengono poi codificate l'anno successivo, sempre in Italia, a Stresa, dando una netta percezione di quanto l'Europa nasca con dinamiche interconnesse a una Nazione che ne è protagonista che è stata protagonista nella sua fondazione e che dovrà essere protagonista anche nel riportare un'attenzione strategica su quei temi che la videro nascere. Quando faccio riferimento ai Trattati di Roma, faccio riferimento non tanto ai primi 37 articoli, che evidentemente delineano i principi secondo i quali alcune Nazioni, a dodici anni da un terribile conflitto come la Seconda guerra mondiale ritenevano utile e conveniente mettersi insieme, ma all'articolo 38 e seguenti, quando, entrando nel merito, scelsero l'elemento su cui creare un modello economico forte e prospero. Erano persone che avevano avuto vittime in famiglia, che avevano avuto terribili esperienze solo dodici anni prima. A ben guardare, la nostra memoria sembra molto prossima, quando immaginiamo che cosa facevamo dodici anni fa. Ebbene, immaginiamo quelle sei Nazioni che scelgono, attraverso i Padri fondatori dell'Europa, di convergere su un obiettivo comune. Maggiore prosperità per il popolo tedesco, per il popolo italiano, per il popolo francese, per il popolo belga, per quello olandese, per quello lussemburghese, in un'ottica, però, di aggregazione che doveva venire. Qual era il pilastro su cui l'Europa converge? L'industria? No, perché l'industria, nonostante si andasse verso la crescita di quel settore di natura economica, sceglie di adottare un altro tipo di principio. È l'agricoltura. L'agricoltura è il pilastro fondamentale su cui si costruisce un modello d'Europa a garanzia della sicurezza alimentare e a garanzia della manutenzione del territorio. L'agricoltore è fondamentale nella gestione del territorio. L'agricoltore era, per i Padri fondatori d'Europa, il centro della tenuta del nostro sistema, anche dal punto di vista ambientale, oltre che dal punto di vista dell'approvvigionamento del cibo, che era evidentemente mancato nella fase del conflitto più di ogni altra cosa. Nel tempo, l'Europa questo lo ha considerato un elemento secondario, sempre di più. La centralità che si era persa, oggi, con il nostro Governo viene ritrovata anche in quel consesso. Il 21 marzo si torna a parlare tra *leader* europei, dopo decenni, della agricoltura come questione centrale da affrontare a fianco dei grandi conflitti ai quali spesso è interconnessa. Lo dico perché, se si contesta la visione strategica, si deve comprendere la ragione per la quale noi riteniamo l'agricoltura un elemento eccezionalmente importante; insieme alla pesca, un elemento di garanzia per la produzione agroalimentare, per la tenuta del nostro sistema di approvvigionamento e anche quindi per rendere l'Europa protetta e l'Italia protetta da ogni rischio di condizionamento, anche attraverso le catene alimentari, e per la nostra libertà in futuro. Su questo abbiamo incentrato la nostra azione, fin dall'inizio, con un aumento esponenziale dei finanziamenti, con la revisione del PNRR, raddoppiando le cifre che erano indirizzate al rafforzamento del sistema agricolo, alla produzione di energia solare, che ha visto protagonista il Ministero dell'agricoltura con il finanziamento, per ora, di 13.500 aziende che produrranno energia pulita senza sottrarre neanche un metro di terra a quello per cui la terra è finalizzata: la produzione di cibo. Abbiamo avuto modo di proteggere il nostro sistema. Lo abbiamo fatto, anche se non tutti erano d'accordo, con una norma che incide sul nostro modello di produzione che, a nostro avviso, deve essere legato alla terra, al lavoro, alla alla qualità come elemento portante. Per noi, per la nostra tradizione, il cibo non è solamente un elemento nutrizionale, ma è anche un elemento di carattere culturale, identitario, di benessere. Per questo abbiamo contrastato l'ipotesi della produzione di cibo coltivato in laboratorio. Lo abbiamo fatto in Italia. Abbiamo valutato positivamente il dibattito che ne è emerso e abbiamo valutato altrettanto positivamente che in Europa tante altre nazioni hanno sottoscritto il documento presentato da Italia, Francia e Austria, che considera questa produzione un potenziale pericolo per la salute, per l'ambiente, per la cultura, per il lavoro, per l'identità, per tutti quei fattori che, in quest'Aula, avevamo denunciato, ascoltando parte del Parlamento rivendicare la possibilità che l'Europa impedisca all'Italia di normare in questo settore. È stato esattamente il contrario. In Europa seguono il buon esempio di una Nazione che di qualità ne sa evidentemente, ai loro occhi, spesso più di loro. Anche dall'altra parte dell'oceano, la Florida ha scelto di seguire l'esempio dell'Italia, con una normativa di questo tipo e tanti altri Stati stanno discutendo dell'argomento. Purtroppo, noi interveniamo in un settore che nel tempo è stato marginalizzato. L'agricoltore è stato letto come problematico per l'ambiente; non il primo custode dell'ambiente, ma un problema per l'ambiente. Il tentativo è stato quello di trasformare la PAC in uno strumento pedagogico educativo dell'agricoltore, piuttosto che in uno strumento che incentiva la produzione, che dà la possibilità all'agricoltore di garantirsi il reddito a prescindere dal valore dei suoi prodotti, per il suo ruolo che veniva considerato fondamentale da chi ha immaginato lo strumento di custode di alcune aree. Col senno di poi abbiamo verificato, immagino tutti, che ciò corrisponde esattamente a una visione strategica che i Padri fondatori dell'Europa avevano chiara all'epoca…

lo stanziamento delle spese e la loro finalizzazione. La questione secondo me più rilevante è la visione strategica del Paese, provando a coniugare gli interventi del Parlamento in una visione di rilancio dell'*asset* primario. Purtroppo,

Il Parlamento ha migliorato ulteriormente questo intervento, dando la possibilità di intervenire anche con una moratoria per le imprese che hanno una diminuzione delle produzioni del 30 per cento, in maniera da anticipare il problema rispetto anche all'anno che verrà.

20 miliardi l'intervento in favore dell'agroindustria e del settore agricolo e ciò permetterà ulteriormente di avere disponibilità in questo senso. Abbiamo lavorato per garantire al mondo agricolo

quegli imprenditori agricoli, che desidero salutare e ringraziare non tanto per quello che hanno fatto prima dell'alluvione, ma per quello che hanno fatto dopo, con coraggio, ricostruendo e restando al loro posto, cercando di tenere in piedi quell'attività. A loro dobbiamo tanto ed è anche per questo che abbiamo cercato risorse in ogni modo, per andar loro incontro. *(Applausi)*. Siamo intervenuti su alcune fitopatie molto rilevanti. Certo, anche in quel caso si può fare di più, si può fare tutto, ma le condizioni nelle quali ci siamo trovati, con le criticità che ben conoscete dal punto di vista dell'economia dello Stato, ci permettono di fare sempre un passo alla volta per non creare illusioni. Siamo comunque intervenuti su filiere delicatissime, come quella del kiwi che per alcune aree del Paese è strategica, quella delle pere e ovviamente vite. Siamo stati colpiti dalla peronospora, quest'anno in maniera più significativa rispetto agli anni precedenti; abbiamo fatto un primo intervento di 7 milioni, che è stato insufficiente, poi abbiamo stanziato altri 10 milioni, altri 30 milioni li metteremo ora e continueremo ad intervenire man mano che troveremo risorse. *(Applausi)*.

per una legge che doveva aumentare il numero di assicurati diminuendo i premi assicurativi e che, invece, ha diminuito il numero degli assicurati, aumentando i premi assicurativi e di questo forse qualcuno del passato è responsabile. *(Applausi)*. Abbiamo lavorato sulla trasparenza dei prezzi di mercato. Ha ragione lei, senatore Bergesio: non siamo intenzionati a intervenire in maniera impropria sull'impresa e sulla libertà di impresa. *(Applausi)*. che non ci debba essere, come è normale, una posizione dominante che mette in ginocchio gli agricoltori. Se allora è impraticabile la scelta di imporre un prezzo di vendita all'imprenditore agricolo, noi controlleremo tutti quelli che invece compreranno compreranno prodotti a un prezzo che sia inferiore al costo medio di produzione. *(Applausi)*. Il che significa utilizzare al meglio le nostre Forze dell'ordine, cercando, ovviamente nella libertà di impresa, di punire chi eventualmente viola le regole della concorrenza leale. Su questo abbiamo lavorato. Qualcuno parlò di pioggia di posti di lavoro al Ministero, ebbene assumeremo più carabinieri, più ispettori del controllo qualità e repressioni frodi *(Applausi)* perché il pubblico impiego non è un posto per raccomandati, ma quando funziona quando funziona bene è un luogo in cui la burocrazia, quando fa il suo lavoro, aiuta il sistema a funzionare meglio e a rispettare le regole, quindi sono contento che si stia andando in questo senso. Abbiamo per questo anche rafforzato uno strumento, Ismea, del quale spesso ci si è riempita la bocca. Ismea è tornata ad essere centrale per per arrivare non solo all'analisi da pubblicare nei telegiornali e sulle statistiche, ma anche ad intervenire in modo attivo sulle verifiche, come quella che ho appena citato, in correlazione con le Forze dell'ordine. Abbiamo lavorato sui pannelli fotovoltaici. fotovoltaici. Ho rivendicato il fatto che abbiamo, da una parte, triplicato la previsione di produzione di energia solare che era stata fatta dal Governo precedente, e dall'altra abbiamo posto fine a uno scempio uno scempio che anche questo Parlamento nel 2021 sentì come un'emergenza, normando e dicendo che bisognava individuare le aree idonee per le installazioni di pannelli. *(Applausi)*. Dopo quattro anni, però, visto che non si riusciva a fare per responsabilità di tutti, l'abbiamo fatto senza guardare in faccia a nessuno, senza guardare in faccia alle *lobby*, agli articoli, a quelli che ti attaccano perché hai posto un freno all'aggressione ai terreni agricoli che sono definiti così per produrre per produrre cibo, per produrre nutrimento. Se vuoi produrre sul tuo terreno altro, senza il rispetto della vocazione che permette anche interventi di fiscalità agevolata,

è una delle criticità maggiori che stiamo affrontando, come la sta affrontando il resto del mondo, perché la peste suina non è una questione italiana. Lo stiamo facendo - ha ragione il senatore De Carlo - spesso in maniera più attenta anche di altre Nazioni e questo ci viene riconosciuto. Abbiamo, a questo scopo, schierato anche l'Esercito. Qualcuno ha detto che l'Esercito deve fare altro, ma io penso che l'Esercito possa essere tranquillamente utilizzato e anzi ci auguriamo che venga utilizzato più per questioni di questa natura che per altro quando si rende disponibile, come è avvenuto, e ringrazio il ministro della difesa Crosetto e tutto lo Stato maggiore per aver garantito la possibilità di utilizzare nel contrasto al primo veicolo che c'è oggi di diffusione della peste suina che è l'ungulato, anche l'Esercito, non riuscendo a farlo in maniera efficace con il solo aiuto di chi è abilitato all'uso delle armi. Anche su questa vicenda dell'abbattimento degli ungulati in Italia per la scienza, non per il Ministro, in un quantitativo eccessivo rispetto a quanto sia tollerabile dall'equilibrio del nostro ecosistema, abbiamo anche aumentato di un mese la possibilità di attività venatoria rispetto agli ungulati e anche l'utilizzo dei visori notturni che ci sono stati segnalati come elementi che possono aiutare ad affrontare e a risolvere questo problema. non è un decreto per l'attività venatoria e quindi, rispetto alle polemiche, mi assumo la responsabilità di dire con serenità che avremo altre occasioni per discutere nel merito dell'attività venatoria, del contrasto a chi impedisce attività lecite in questo Stato, ma non è questo il decreto per farlo. Siamo andati incontro quindi agli inviti e alle sollecitazioni a ridurre il tema dell'attività venatoria solo connessa alla peste suina africana e non invece incidente su

ne abbia stabilito le modalità di attuazione. Così siamo intervenuti su altre due criticità, la brucellosi e la tubercolosi bovina. Il commissario ulteriore che è stato istituito avrà una serie di puntualizzazioni, anche grazie al Parlamento, per interventi che non stabilizzino

È stato Considerato dalla FAO e dalla CEE, allora l'Unione europea si chiamava così, non più specie aliena, perché era ormai endemica nel Mediterraneo. Eppure nessuno ha pensato a prevedere che ci potesse essere una fluttuazione di abbondanza come quella che c'è stata nella scorsa stagione. Siamo intervenuti immediatamente su due pilastri: in primo luogo abbiamo cercato di arginare la presenza di un crostaceo che è un pericolo per l'ambiente pericolo per l'ambiente e purtroppo anche per alcune attività come la venericoltura che è stata messa in ginocchio. La mia solidarietà totale è andata ai nostri pescatori

avremo la possibilità di nominare un commissario che dovrà affrontare in termini contingenti la criticità nel settore della venericoltura, ma anche e soprattutto il processo di diminuzione della presenza di questa specie

il granchio blu è un alimento molto apprezzato e dal grande valore di mercato in tante altre Nazioni. Anche da questo punto di vista gli interventi che abbiamo fatto sembrano aver avuto dei ritorni in termini occupazionali. Abbiamo lavorato sulle razze autoctone e sulla difesa di alcune razze che rischiano in Italia un indebolimento. Abbiamo lavorato - e ringrazio il senatore La Pietra ancora una volta - su Granaio Italia, un'altra questione che era stata lasciata inevasa, rinviata ogni anno.

immaginare di stabilizzare la Xylella con devoluzioni infinite, senza avere una strategia che possa mettere in condizione o di reimpiantare

impossibilitati a produrre buon olio in Puglia. Su questo abbiamo investito risorse che serviranno esattamente al tema. Così come siamo intervenuti sul bostrico, altra criticità che riguarda il nostro patrimonio boschivo e forestale. boschivo e forestale. Ha ragione chi crede come noi nella scienza. È chiaro che noi non vogliamo mutare il nostro modello e le tecnologie evolutive avanzate sono una risposta in linea con lo sviluppo che la natura farebbe, anche probabilmente probabilmente in assenza dell'uomo, ma per il quale ci vorrebbe troppo tempo. Cerchiamo di avere un insieme di piante che siano meno idroesigenti, più produttive e in linea con quello che la scienza in Italia - con quello che Nazareno Strampelli, in particolare - con l'ibridazione, è già riuscita a realizzare nel tempo. Non ci fermeranno gli ecoterroristi con la distruzione dei campi sperimentali. Chi contrasta la scienza con attentati si chiama terrorista. Non ci sono altri termini per definirlo. *(Applausi)*. Si vuole infatti creare terrore intorno a un argomento serio come quello di cui parliamo. Si può discutere, ma non bisogna usare nessun atto di violenza, anche quelli di questo tipo. Per questo lavoriamo sulla proroga e lavoriamo in Europa per convincere le Nazioni che non hanno lo stesso tipo di approccio che abbiamo noi su questa strada. Poi c'è una diminuzione dei costi. Di solito le poltrone vengono moltiplicate, ma nel nostro Governo e nel nostro Ministero le abbiamo diminuite. Abbiamo diminuito i consigli di amministrazione, abbiamo cancellato alcune società che nel tempo avevano visto solo aumentare i costi di gestione. Una di queste era SIN alimentare e delle foreste*. Avremo modo di confrontarci su quello che è successo in quello strumento in questi anni, ma non c'è ragione di farlo durante una decretazione che invece ci vede, in linea con la tutela dei lavoratori dell'azienda stessa, garantire una diminuzione dei consigli di amministrazione, una diminuzione di spesa e un aumento di efficienza, che è ciò a cui miriamo. Mi scuso, presidente La Russa. Mi ha lasciato terminare, nonostante avessi superato i tempi. Ringrazio per la pazienza. PRESIDENTE. Non li ha ancora superati. Ha ancora cinquanta secondi. Ovviamente mi auguro che qui e nell'altro ramo del Parlamento ci possa essere un atteggiamento in linea con quella che è stata fin dall'inizio la vocazione di confronto con tutte le forze politiche e con i colleghi che mi hanno preceduto (Stefano Patuanelli, De Castro)

che facevano già parte di un disegno di legge precedente alla tragica fine di Satnam, con la conseguenza rispetto a un atto criminoso. nuovo che un criminale è un criminale e un imprenditore agricolo è un'altra cosa. Io credo che colui che ha compiuto quell'atto scellerato sia un criminale e che chiamarlo imprenditore agricolo sia fuorviante, perché gente come lui deve stare lontano da qualsiasi consesso sociale, possibilmente in galera. Ha parlato esattamente trenta minuti, che è il termine massimo che, a discrezione del Presidente, può essere concesso a una replica di un componente del Governo, quindi nel pieno rispetto del Regolamento. Lo dico per il collega

a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1138, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per portare oggi in Senato e riflettere su quanto accaduto lo scorso *weekend* a Milano. Durante il punto stampa della segretaria del Partito Democratico Elli Schlein, dentro al Pride, quattro giornalisti sono stati molestati da un uomo che ripetutamente li ha palpeggiati e toccati nelle parti intime. Innanzitutto è importante riflettere su come tale manifestazione, che dovrebbe essere dedicata alla celebrazione dei diritti e dell'inclusività, si possa trasformare in occasione di abuso e prevaricazione. Ci saremmo aspettati una risposta da parte degli organizzatori dell'evento, che invece tarda ad arrivare. Le molestie - ricordo - rappresentano un attacco alla dignità di chi le subisce.

Gli autori delle violenze contro gli uomini sono esattamente gli stessi uomini, per la maggior parte; anche su questo potremmo fare una riflessione. Vorrei intanto esprimere la mia vicinanza e solidarietà a Chiara Daffini e ai suoi colleghi. È doveroso sottolineare che la gravità dell'accaduto non viene minimamente attenuata dal fatto che tra le vittime ci siano degli uomini, poiché la violenza, la molestia e l'abuso non conoscono sesso e devono essere condannate con la stessa fermezza e la stessa determinazione in ogni circostanza e senza distinzione di genere. Ci tengo a ribadirlo anche in quest'Aula, perché questo episodio è passato molto in sordina. Non ho sentito ad esempio le reazioni feroci delle femministe, sempre pronte a urlare e a tuonare indignazione. Non ho visto le levate di scudi dei tanti giornalai di sinistra né dei tanti *blogger* travolti dalla passione dei diritti civili. Laddove in altri contesti la sinistra avrebbe proposto interrogazioni, ispezioni e dispensato pubblici anatemi verso una società patriarcale che uccide l'uguaglianza, qui arriva il corto circuito del silenzio. A mio avviso, non si può risolvere una molestia sessuale solo con un lieve disappunto e francamente da una manifestazione definita per antonomasia quella dei diritti ci saremmo aspettati di più, almeno una parola in più.

Oggi siamo al 3 luglio e credo che mi dovrò rivolgere, dopo aver provato due volte con il Senato, direttamente alla dottoressa Sciarelli perché dedichi una puntata di «Chi l'ha visto?» alla mia interrogazione, visto che il ministro Urso non risponde. Si tratta della disgregazione di Confindustria Moda, l'associazione delle associazioni del settore della filiera della moda, del tessile, del lusso, degli accessori, che sotto lo sguardo del Ministro si sta dissolvendo. Volevo pertanto sapere dal Ministro se ne fosse a conoscenza e se stesse esercitando la sua *moral suasion* per fare in modo che Confindustria Moda, una entità una entità che serviva a fare sistema in un settore importantissimo del *made in Italy* e delle nostre esportazioni, non si disgregasse. Purtroppo gli ho posto tali quesiti il 25 gennaio ed è la seconda volta che sollecito.

del Senato possano parlare con l'ufficio rapporti con il Parlamento del Ministero del ministro Urso perché finalmente mi risponda.

proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"